senatrice Zedda, legge di bilancio per l'anno 2023-2025, è stato presentato in data 23 marzo 2023, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati e trasmesso al Senato il 12 luglio 2023. Il disegno di legge in esame, modificato in sede referente dalla 6a Commissione del Senato, consta di 23 articoli, distribuiti in cinque titoli. Negli articoli dall'1 al 4 troviamo i principi generali e la riforma dello statuto del contribuente: questi compongono il titolo I. Agli articoli 1-3, il titolo I contiene i principi generali e i tempi di esercizio della delega. All'articolo 4 troviamo i principi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con particolare riguardo alla disciplina dell'interpello. Andando nel particolare, l'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, indicando i principi e i criteri direttivi generali e specifici cui deve attenersi la stessa (comma 1), disciplinando le modalità e i termini di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativi (commi 2 e 3) e il meccanismo di slittamento del

particolare per gli atti di trasferimento o di destinazione di beni e diritti in favore di persone con disabilità e l'applicazione dei principi e criteri direttivi generali di cui alla legge sul federalismo fiscale. Nel corso dell'esame in sede referente al Senato si attribuisce al Governo, nella predisposizione dei decreti delegati, il compito di assicurare la piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali, di cui alla legge sul federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n. 42), al decreto legislativo n. 68 del 2011, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province e per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome. L'articolo 3 reca i principi e i criteri direttivi di delega per la riforma del sistema fiscale, con riguardo agli aspetti internazionali e sovranazionali del sistema tributario, con particolare riferimento all'adeguamento dell'ordinamento tributario nazionale agli *standard* di protezione dei diritti stabiliti dal diritto dell'Unione europea. L'articolo 4 stabilisce che il Governo, nell'esercizio della delega per la revisione del sistema fiscale, osservi una serie di principi e criteri direttivi per la revisione dello statuto dei dei diritti del contribuente, tra i quali, oltre al rafforzamento dell'obbligo di motivazione degli atti impositivi e alla valorizzazione dei principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto, rilevano specialmente i principi introdotti in materia di interpelli. Il titolo II, che va dall'articolo 5 all'articolo 15, riguarda i tributi, rappresenta la parte più ampia della delega ed è articolata in tre capi: al capo I, agli articoli da 5 a 8, troviamo le imposte sui redditi, IVA e Irap e l'articolo 9 nel quale confluiscono ulteriori disposizioni sulla materia. Al capo II, agli articoli dal 10 al 12, troviamo tutte le altre imposte indirette. Al capo III, articoli dal 13 al 14, troviamo i tributi regionali e locali. Al capo IV troviamo l'articolo 15 concernente la disciplina dei giochi. Nello specifico, l'articolo 5 contiene i principi e criteri direttivi in materia di Irpef. In termini generali si dispone la revisione e la graduale riduzione dell'Irpef, nel rispetto del principio di progressività e tendenzialmente e gradualmente diretto al raggiungimento di un'aliquota unica. Nel riordino delle agevolazioni si deve tener conto delle relative relative finalità, con particolare riguardo ad alcuni elementi. Si prevede inoltre il graduale proseguimento dell'equità orizzontale attraverso, tra l'altro: l'applicazione della stessa area di esenzione fiscale e dello stesso carico impositivo Irpef, indipendentemente dalla natura del reddito prodotto e la possibilità del contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori. Specifici principi sono previsti per i redditi agrari, con l'obiettivo di favorire ed agevolare l'aggiornamento delle classi e qualità di coltura, prevedendo tra l'altro un regime di favore per i redditi ottenuti da soggetti titolari di pensione e di redditi modesti che svolgono attività agricole. Per quanto concerne i redditi da fabbricati, il disegno di legge indica la possibilità di estendere il regime della cedolare secca agli immobili adibiti ad uso diverso da quello adibito qualora - è stato precisato nel corso dell'esame presso la Camera - il conduttore sia un esercente, un'attività d'impresa di arti o di professioni. Diversi principi e criteri direttivi concernono i redditi di natura finanziaria, rispetto ai quali si prevede la creazione di un'unica categoria reddituale, determinando il valore di tali redditi sulla base del principio di cassa, assicurando una più ampia possibilità di compensazione

Per quanto riguarda il lavoro autonomo e nell'ottica di semplificazione e razionalizzazione, si prevede in particolare il concorso alla formazione del reddito di tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo conseguiti, l'allineamento del trattamento fiscale degli immobili strumentali nonché di quelli ad uso promiscuo, la riduzione delle ritenute operate sui compensi nel

al regime dell'imposta sul reddito della società e l'assoggettamento ad aliquota proporzionale allineata a quella ordinata dall'Ires. Sono infine contemplati specifici interventi sui cosiddetti redditi diversi. L'articolo 6 reca i princìpi e i criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti. In sintesi si prevede, oltre alla semplificazione dell'allineamento tra valori civilistici e fiscali, un doppio regime agevolato rispetto all'Ires ordinaria: accanto all'aliquota ordinaria (attualmente pari al 24 per cento), infatti, in sostituzione

L'articolo 7 reca i principi e i criteri direttivi specifici per la revisione dell'Iva prevedendo una ridefinizione dei presupposti dell'imposta in modo da renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea, la revisione della disciplina delle operazioni esenti, la razionalizzazione del numero

diversi ambiti specifici attinenti all'imposizione sui redditi, tra i quali si colloca innanzitutto la razionalizzazione e la semplificazione dei criteri di determinazione del reddito d'impresa prevedendo inoltre la razionalizzazione degli incentivi alle imprese e della fiscalità di vantaggio; sono stabiliti principi e criteri direttivi con riferimento ai redditi delle imprese che accedono agli istituti disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, alle società "di comodo", nonché con riferimento ai regimi agevolativi per gli enti del terzo settore e alle misure fiscali per gli enti sportivi. L'articolo 10 specifica i principi e i criteri direttivi specifici relativi ai tributi indiretti diversi dall'Iva, con particolare riferimento all'imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni e imposta di bollo. L'articolo 11 reca i principi e i criteri direttivi specifici a cui il Governo è tenuto ad attenersi per la revisione revisione della disciplina doganale, attraverso il riassetto del quadro normativo in materia doganale, il completamento della telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali, il potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli ed il riordino delle procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione. L'articolo 12 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega L'articolo 12 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento alle accise e alle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Si prevedono vari principi e criteri direttivi tra i quali la rimodulazione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica e sul teleriscaldamento in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto. L'articolo 14, introdotto al Senato, stabilisce principi e criteri direttivi specifici volti a realizzare una revisione del sistema fiscale degli enti locali attraverso un consolidamento dell'autonomia finanziaria; la piena attuazione del federalismo fiscale, una razionalizzazione dei tributi e una modernizzazione del sistema di rilevazione dei dati volta a ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale. L'articolo 15, contenente i principi e i criteri direttivi in materia di giochi, conferma innanzitutto il modello organizzativo del sistema dei giochi basato sul regime concessorio e autorizzatorio. Reca inoltre i principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici.

un ordigno ad altissimo potenziale esplose nella sala d'attesa della stazione di Bologna, causando 85 vittime e oltre 200 feriti. Quelle immagini drammatiche di devastazione, di sangue e di disperazione sono ancora oggi scolpite nel profondo della nostra memoria; immagini che non dobbiamo e non vogliamo dimenticare perché la memoria è il collante della nostra identità. Nulla è più vigliacco e nemico della civiltà di un attentato fatto da chi proditoriamente, nascondendo la mano, colpisce cittadini innocenti, uomini, donne e bambini, che quel giorno cercavano un inizio di estate, magari felice, e hanno trovato invece una ingiusta morte. Tramandare la memoria affinché non venga mai meno l'amore per quei valori di libertà e democrazia che sono scolpiti nella nostra Costituzione è un impegno che non possiamo, non vogliamo e non dobbiamo trascurare. Un impegno di verità e conoscenza che dobbiamo a tutte le vittime del terrorismo, in relazione al quale ritengo fondamentale proseguire anche in questa legislatura l'importante opera di desecretazione degli atti delle Commissioni parlamentari d'inchiesta, che hanno indagato su molte tragiche pagine del nostro passato, al fine di rimuovere ogni ombra, ogni dubbio e ogni interrogativo ancora aperto. Va doverosamente ricordata la definitiva verità giudiziaria che ha attribuito alla matrice neofascista la responsabilità di questa strage. Desidero inoltre rivolgere un pensiero alle associazioni dei familiari delle vittime delle stragi e del terrorismo che ringrazio per l'instancabile opera di sensibilizzazione. In questa giornata, che è una giornata di memoria, ma anche di dolore e di condivisione, è però importante ricordare l'orgoglio, il coraggio e la determinazione con cui tutta la Nazione non si è mai - ripeto mai - piegata al ricatto della paura e, unita, ha sconfitto il terrorismo, contrapponendo alla barbara violenza delle bombe la forza della giustizia e della democrazia. Nel rinnovare ai familiari delle vittime della strage di Bologna e di tutte le vittime del terrorismo, nessuna esclusa, la mia profonda e sincera vicinanza e il mio commosso pensiero, invito l'Assemblea, esattamente nel momento in cui nel 1980 quella tragica bomba esplodeva a Bologna, a osservare un minuto di silenzio.

Dichiaro

stiamo imboccando la strada giusta, la strada della semplificazione, della razionalizzazione degli adempimenti, delle maggiori garanzie per i cittadini per un miglior contraddittorio, diritto d'accesso, autotutela e gradualità dei versamenti, per il raggiungimento della strada della collaborazione, della fiducia e della maggiore chiarezza. Una delega del resto che non mi pare abbia ricevuto particolari critiche dagli osservatori del settore o dagli operatori, dai tributaristi e dagli operatori, dai tributaristi e da chi davvero conosce il settore del fisco, a parte la CGIL, che non mi sembra una nota organizzazione di fiscalisti e tributaristi o a parte le "renzate" che inventano prelievi forzosi inesistenti. *(Applausi)*. D'altronde siamo un po' abituati alle renzate: abbiamo scoperto che Renzi

onora più che altro il lavoro e il sacrificio di tanti cittadini italiani, l'impegno con cui tanti cittadini italiani cercano di avere un rapporto positivo col fisco, fisco, il sudore di chi si alza alle 4 del mattino, solleva una saracinesca e sa che tutti gli anni deve lavorare almeno per metà dell'anno per pagare le tasse. tasse. D'altro canto, non tutti abbiamo la fortuna di lavorare per società del lusso con sede in Delaware, non tutti abbiamo la fortuna di trovare fortuna di trovare dei soldi nella cuccia del cane, non tutti abbiamo la fortuna di avere commesse milionarie vendendo armi *(Applausi)*. Questo non è il quadro degli italiani: gli italiani sono persone che cercano di portare avanti la loro piccola impresa. Bisogna anche interrompere una falsa rappresentazione per la quale chiunque non paghi le tasse è un evasore e quella per cui chiunque non paghi le tasse è un lavoratore autonomo.

chi ha commesso errori formali nella compilazione della modulistica, ma non ha il dolo di aver voluto evadere le tasse e quando gli arriva la cartella la paga, non è un evasore; chi chi riceve una cartella dall'Agenzia delle entrate non è automaticamente un evasore, perché sarebbe come dire che chi è indagato dalla procura della Repubblica è automaticamente un criminale. *(Applausi)*. Sono

o anche perché l'Agenzia delle entrate, che ha fatto degli accertamenti che erano legittimi per il recupero dell'evasione ma non erano fondati, poi vince il contenzioso. Dico questo perché lo spirito con il quale ho depositato il mio ordine del giorno va in questa direzione: nessuno vuole che ci sia più evasione e nessuno è dalla parte degli evasori. Dico anche che

quella fattura non la emette. L'evasione è trasversale in tutti i settori della vita pubblica, purtroppo è una parte del sistema contro cui dobbiamo lottare. Non possiamo poi pensare di recuperare il rapporto col contribuente raccontandogli la favola che paghiamo tutti per pagare meno.

di più, i cittadini italiani hanno pagato di più, ma le tasse sono aumentate. È dunque giusto recuperare un rapporto col fisco che sia equilibrato e l'ordine del giorno che ho presentato e che è stato accolto va anche in questa direzione.

adottano la pratica di continuare ad appellare, anche dopo tanti gradi di giudizio, sentenze che sono loro sfavorevoli. È vero che il 76 per cento dei ricorsi vede la vittoria del fisco, ma è altrettanto vero che ci sono molte persone che magari non fanno ricorso. È altrettanto vero che, per la ragione che ho detto prima, il processo tributario

ha subito un accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate, secondo la quale consumava più acqua delle automobili che dichiarava. Ha portato all'Agenzia delle entrate i dati tecnici del proprio macchinario, dimostrando che consumava più acqua di quelle che aveva preso in considerazione l'Agenzia delle entrate, non c'è stato verso. Ha fatto ricorso alla commissione tributaria, ha vinto il primo grado e ha vinto il secondo grado. La Cassazione ha però annullato con rinvio al primo grado, ha rivinto il primo grado e ha rivinto il secondo grado. Ha chiesto la pace fiscale, perché non ne poteva più, non ne poteva più, ma gli è stata negata, perché non aveva vinto tutti i gradi del giudizio, perché aveva perso in Cassazione e quindi è ancora pendente il giudizio della Cassazione.

da contenziosi tributari che potevano essere risolti magari con attività di *compliance* o con attività che sono previste all'interno di questa delega. Questa è la ragione che ho cristallizzato nell'ordine del giorno

perché ci sono continui ricorsi. È chiaro infatti che il cittadino paga il suo avvocato. Allora credo che, anche rispetto a questo, ci debba essere un maggiore controllo, per rendere meno odioso e recuperare il rapporto tra fisco e contribuente, che consentirebbe, come indica questo disegno di legge delega, di recuperare l'evasione prima che emerga, prima dell'attività dell'Agenzia delle entrate. È anche in questa direzione che vanno le proposte di razionalizzazione delle aliquote e in questa direzione va il disegno una delle ragioni per le quali questa delega credo sarà molto apprezzata. È chiaro che ci sarà un lavoro importante per darle forma, perché poi, quando si entra nel dettaglio, ovviamente tutto diventa più complicato. Quello che credo sia importante, oggi, è recuperare il rapporto di fiducia e una sana collaborazione tra cittadino e fisco, in modo che i cittadini paghino più volentieri il fisco

a volte si trova a pagare sanzioni assurde e spropositate. Io sono reo, in quanto ho ricevuto una cartella esattoriale. Ad esempio, non io personalmente, ma una persona a me vicina aveva dichiarato due metri quadri di casa in meno di quella che

evasione, dove c'è la vera volontà di dichiarare meno per imbrogliare il fisco e dove magari ci sono semplicemente errori dovuti anche a*...

Signor Presidente, approfitto per salutare in Aula il vice ministro Leo e il sottosegretario Freni, con cui abbiamo condiviso, come opposizioni, un percorso di confronto sempre leale da parte nostra in queste settimane. Sono certa che non sfugga loro, così come non sfugge a noi e a nessuno in quest'Aula, quanto sia centrale, per la qualità del patto sociale che regge la nostra democrazia e la nostra Repubblica, la discussione che oggi facciamo intorno ai temi della delega fiscale. Non si tratta di un argomento di natura tecnica, bensì di un argomento fondante il patto sociale tra cittadini e istituzioni e tra categorie di cittadini. È indubbio, infatti, che un sistema fiscale sia la cartina di tornasole della capacità di un Paese e di una democrazia di produrre equità sociale, redistribuzione e parità di condizioni in partenza. È altrettanto indubbio che il nostro sistema abbia bisogno di una profonda revisione per rispondere al dettato costituzionale che ci indica, appunto, equità, giustizia, progressività fiscale e certezza del diritto. Purtroppo per il Paese, la delega che oggi discutiamo si muove in direzione opposta a questi principi. Sui grandi *vulnus* del nostro sistema fiscale (penso alla fuga dall'Irpef di intere categorie di contribuenti, all'evasione *monster* che non appare in altri Paesi europei, all'incertezza e all'arbitrarietà dei rapporti tra il fisco e il contribuente) voi

Il Governo, di fronte a questi temi, sta proponendo ricette inadeguate, se non sbagliate, ispirate all'idea, che noi troviamo gravemente eversiva rispetto al rapporto di fiducia tra cittadini e Stato, che le tasse siano un sopruso, se non addirittura un pizzo estorto dalle istituzioni ai cittadini. Presidente, non è sfuggito all'opinione pubblica e nemmeno a noi, evidentemente, che il percorso di questa delega sia stato costellato da dichiarazioni improprie sui temi fiscali di diversi esponenti del Governo, che quotidianamente hanno ostacolato o orientato, a seconda dei punti di vista, il lavoro del vice ministro Leo, con messaggi esplicitamente riferiti a futuri condoni o a sanatorie, che hanno incoscientemente messo a rischio misure di recupero fiscale che sono tuttora in atto. Penso, in particolare, alla rottamazione *quater*, rispetto al cui *iter* anche il MEF ha fatto trapelare esplicita preoccupazione. In economia, signor Presidente, il Vice Ministro sa e mi può insegnare che le aspettative di norme future sono in grado di produrre effetti sul gettito attuale, reale. Ne abbiamo testimonianza proprio in questi giorni, con i dati che evidenziano un crollo del gettito dell'IVA. È tutto frutto di un percorso che noi abbiamo ritenuto sbagliato, anche nel metodo, improprio e irresponsabile di gestire una delega così delicata. Anziché porre rimedio alla fuga dall'Irpef con il suo corretto sistema di progressività, la delega, da una parte, accentua il carattere frammentario del sistema fiscale, con la proliferazione di regimi sostitutivi e cedolari e, dall'altra, non abbandona l'orizzonte per noi assolutamente iniquo e sbagliato della *flat tax*, un modo per fare parti uguali tra diseguali, quella che, secondo la famosa massima di don Milani, è la peggiore delle ingiustizie.

Proprio per riprendere il tema dell'equità orizzontale, di cui pure la delega parla - anche se ne parla soltanto - se noi oggi confrontassimo diverse categorie di contribuenti a parità di reddito (poniamo 50.000 euro), scopriremmo che un lavoratore dipendente pagherebbe un onere contributivo 1,6 volte più alto di quello di un percettore di dividendi, due volte superiore a quello di chi dà in affitto i propri immobili, ricevuti magari per trasmissione familiare, con la cedolare secca e 2,8 volte maggiore di quello di un professionista in regime forfettario. La diminuzione delle aliquote, che voi indicate come orizzonte della delega, premia anche all'interno di queste categorie i redditi più alti, senza nulla redistribuire a quelli più bassi, mentre noi abbiamo proposto un sistema completamente diverso, con un'aliquota continua, secondo il modello tedesco, più equo, progressivo e consonante con il dettato costituzionale. Come se non bastasse, la delega contribuisce a questa ingiustizia, guardandosi bene dal ridurre i regimi di tassazione separata o cedolare, ma, al contrario, aggiungendone altri. Penso, in particolare, all'estensione della cedolare secca agli immobili strumentali: da ex amministratrice locale che ha gestito per tanti anni una delega delicata come quella del commercio in una grande città come Milano, questa misura mi risulta particolarmente incomprensibile e odiosa per due ordini di ragioni. La prima ha a che fare proprio con l'equità e la vitalità del sistema del commercio di vicinato e di prossimità; l'altra ha che fare con la riduzione della base imponibile per le addizionali comunali e regionali. Signor Presidente, signor Vice Ministro, le nostre città hanno bisogno di mantenere accese le luci dei piccoli commercianti, degli artigiani e degli operatori economici di prossimità e di vicinato, che oggi sono strozzati da affitti troppo alti per i loro negozi e i loro immobili, che spesso chiudono per questa ragione. *(Applausi)*. La misura che voi proponete va tutta a vantaggio dei proprietari immobiliari e niente ridistribuisce o condivide con i piccoli operatori che rendono vive le nostre città e risulta del tutto incomprensibile perché abbiate rigettato la nostra proposta emendativa su questo tema. tema. In conclusione, vengo a un altro aspetto estremamente critico dell'impostazione della delega. L'insieme delle misure previste, compresa quella sulla cedolare secca, contribuiscono al risultato di ridurre il gettito per enti locali e Regioni, soggetti erogatori di servizi essenziali per i cittadini, che rischiano di dover sostenere il peso di questi servizi con risorse proprie o, peggio, con nuove tasse a livello locale. E nemmeno può bastare a rimediare al danno l'approvazione dell'emendamento da noi proposto, che provava e prova a salvaguardare la finanza degli enti locali, secondo i suggerimenti giunti da ANCI e UPI attraverso la Conferenza unificata, mentre resta assai grave - come altri ribadiranno dopo di me - la bocciatura del nostro emendamento sulla fiscalità delle Regioni, che molto dice dell'*impasse* in cui il Governo si è infilato in materia di autonomia differenziata. differenziata. Infine, non si può tacere su come la maggioranza in Commissione abbia notevolmente peggiorato la disciplina proposta dal Governo in materia di riscossione. Nel nostro Paese l'evasione - non lo devo ricordare al Vice Ministro in quest'Aula - sfiora annualmente i 100 miliardi di euro, anno più anno meno. Abbiamo una propensione all'evasione dell'Irpef da parte del lavoro autonomo e di impresa vicino al 70 per cento; l'IVA è più evasa solo in quattro Paesi dell'area europea. Eppure, oltre ai pessimi segnali che abbiamo richiamato, gli emendamenti approvati dalla maggioranza in Commissione prevedono incomprensibili scudi penali per le dichiarazioni infedeli e sconti per gli evasori. Quale messaggio state dando al Paese, ma anche all'Europa, su un tema che ci vede costantemente sotto osservazione anche dai nostri *partner* europei a livello internazionale? Presidente, non posso fare a meno di rilevare in questa sede, in questi giorni in cui centinaia di famiglie hanno perso il sussidio contro la povertà di poche centinaia di migliaia di euro attraverso un irridente SMS, il doppiopesismo con cui il Governo tratta i poveri e chi ha sbagliato o ha voluto sbagliare nella compilazione della dichiarazione dei redditi il guanto di velluto per chi sottrae risorse alla collettività e il pugno di ferro verso i più bisognosi e i più poveri. Se non vi fosse solo una questione di equità e di giustizia, vi sarebbe comunque un grave tema di sostenibilità per le finanze dello Stato. La Ragioneria generale dello Stato ha già manifestato la sua preoccupazione sulle coperture di questo provvedimento. Facciamo nostra questa preoccupazione, in un momento in cui la crescita del Paese - com'è noto - non è quella che ci saremmo aspettati o avremmo desiderato. Io sono certa che questo argomento troverà sensibile il vice ministro Leo, che è anche guardiano dei conti e della sostenibilità dello Stato, oltre che promotore di questa delega. Quindi, Presidente, spero ci siano le condizioni e la possibilità di tornare su questi temi alle Camere, come noi abbiamo chiesto in altri emendamenti, perché vigileremo su equità e su sostenibilità del provvedimento.

attesa, mantenendo così fede agli impegni presi con gli italiani. La riforma fiscale è necessaria per porre rimedio al difetto del nostro modello tributario, una pressione impositiva fra le più alte delle Nazioni OCSE, un sistema sanzionatorio sproporzionato, complessità e incertezze normative. Il nostro sistema tributario, d'altronde, risale all'epocale riforma degli anni Settanta, alla legge delega n. 825 del 1971. I successivi interventi hanno introdotto elementi di novità, ma senza la sistematicità di una vera riforma (il governo Prodi nel 1997, il governo Berlusconi nel 2003 e il governo Renzi nel 2014). In mezzo a tutto ciò si è collocata una pletora di misure di dettaglio e di interventi affastellati, che hanno reso più complesso il nostro sistema tributario, poi con interventi suppletivi della giurisprudenza. La riforma del sistema fiscale costituisce un elemento chiave del programma di questo Governo, volto al rilancio strutturale dell'Italia sul piano economico e sociale. Il disegno di legge individua fra i principali obiettivi di carattere generale l'impulso alla crescita economica e alla natalità, mediante la riduzione del carico fiscale, l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e l'individuazione di meccanismi fiscali di sostegno a famiglie, lavoratori e imprese. misure necessarie, da un lato, a semplificare, la giungla normativa italiana, incubo di contribuenti ed operatori del settore, e, dall'altro, a modernizzare ed efficientare il comparto fiscale, contribuendo a ristabilire un corretto e positivo rapporto fra Stato e e cittadino, tra fisco e contribuente. Ritengo inoltre di dover sottolineare come questa riforma dia inizio a un'inversione copernicana del rapporto fra Stato e impresa, eliminando l'impostazione ideologica propria di molti Esecutivi precedenti, che vedevano nelle imprese e nel professionista soggetti portati naturalmente

Questo disegno di legge delega si concentra su tre direttrici fondamentali: la certezza del diritto, la semplificazione del sistema e la lotta all'evasione. Quante sono state le modifiche normative? Più di 1.200 in tema di imposte sui redditi e solo 500 in materia di IVA. Abbiamo poi il tema importante dell'International accounting standards board, che viene comunque rispettato. Non tocchiamo principi contabili, ma intendiamo dare regole certe al loro utilizzo. Sul versante internazionale, vi è l'adeguamento delle norme interne alla giurisprudenza comunitaria, all'OCSE, al fine di attirare nuovi investimenti esteri e quindi svolgere il famoso *reshoring*, tutto con lo scopo di portare in tempi rapidi un quadro normativo più chiaro ed omogeneo testi unici con l'obiettivo, tanto anelato, di una codificazione di tutta la materia tributaria. La seconda direttrice sulla quale si è lavorato e si lavorerà è la semplificazione.

in quanto i vari modelli sono composti da 140 pagine del 730, 350 pagine del modello dei redditi delle persone fisiche, 250 pagine del modello dei redditi delle società di persone e 300 pagine del modello dei redditi delle società di capitali. Colleghi,

è sempre rimasto invariato: dagli anni Novanta ad oggi, è sempre oscillato senatore vedo che oscilla la testa, poi ascolterò con interesse il suo intervento, ma questi sono dati inoppugnabili - tra i 75 e 100 miliardi di euro.

l'IVA, l'IRAP. Si prevede una revisione dell'intero meccanismo di tassazione del reddito delle persone fisiche, in modo da raggiungere gradualmente l'obiettivo di un'equità orizzontale attraverso l'individuazione di un'unica fascia di esenzione fiscale e di un medesimo onere impositivo, a prescindere dalle diverse categorie di reddito prodotto, privilegiando in particolare l'equiparazione fra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.

al bilancio - anche in misura forfetizzata, delle spese sostenute per la produzione del reddito di lavoro dipendente e assimilato, nonché la razionalizzazione della disciplina del gruppo IVA, al fine di semplificare le misure previste per l'accesso e l'applicazione. senatori, vorrei anche rivolgere un ringraziamento per il proficuo e concentrato impegno che è stato profuso dai Presidenti e dai relatori delle Commissioni impegnate, che hanno apportato qualificanti innovazioni al testo. Ad esempio, con le forze di opposizione si è ragionato su un'imposta agevolata sui premi di produttività. Con i sindacati si è ragionato sulla revisione della *flat tax* incrementale allineandola alla tredicesima mensilità e agli straordinari. professionista - e qui mi rivesto dei panni di ex amministratrice di un ente locale, perché rammento la forza e la veemenza con le quali imprenditori e professionisti si rivolgevano a noi in quanto consiglieri comunali e amministratori locali e amministratori locali - ossia di non applicare sanzioni o interessi per mancati versamenti su imposte dei redditi regolarmente dichiarati ai soggetti che hanno crediti certificati nei riguardi della pubblica amministrazione per importi pari e fino alla concorrenza del debito d'imposta: è un principio assolutamente fondamentale. Ebbene, noi proseguiremo nella nostra azione all'insegna delle parole d'ordine che abbiamo citato - la certezza, la semplificazione e la lotta all'evasione - tenendo sempre presente che vi sono sicuramente gli equilibri di finanza pubblica da preservare, ma con una direttrice chiara, che è il sostegno alla nostra economia, che vuol dire crescita, sostegno alle famiglie, ai giovani, ai lavoratori e alle imprese; quella crescita è è rivolta anche a un tasso di natalità drammatico, il peggiore dall'Unità d'Italia in poi, pari a 395.000 nati: è bene quindi che tale elemento sia presente in questa legge delega. Agiremo determinati nella direzione della riduzione della pressione pressione fiscale, restituendo sempre maggiore fiducia alla nostra amata Italia.

che la maggioranza si accinge a votare ovviamente parte da un dato, ovvero che non è stato accettato nessun emendamento sostanziale delle opposizioni, ma la cosa più significativa

avete inculcato un ragionamento secondo cui l'Agenzia delle entrate e il fisco intervengono in modo invasivo nei confronti del contribuente.

necessario che vengano pagati i tributi. In questo caso, i tributi, così come prevede la Costituzione, dovrebbe essere pagati in modo proporzionale a seconda del reddito. L'introduzione della *flat tax* è uno schiaffo a questo principio di progressività. Chi più ha, infatti, più dovrebbe contribuire, così dice la Costituzione. Noi invece introduciamo un meccanismo che

di chi può ovviamente farlo. Ripeto invece che i lavoratori dipendenti e i pensionati questa cosa non possono farla, perché sono tassati alla fonte e lo sono in modo superiore a tutte le altre rendite,

ma gli extraprofitti, che sono ovviamente un elemento che in questi anni è aumentato in molte stratificazioni della società, non solo nelle imprese del settore energetico, ma anche

direzione. Vediamo poi anche un altro grande pericolo. Ad esempio, è stato approvato un articolo che considero molto pericoloso da questo punto di vista.

chi contribuirebbe allo Stato a livello centrale. Se infatti ognuno, a seconda delle proprie condizioni, pagherà la propria tassa,

questo? Questo è il dato fondamentale. Le tasse servono per fare i servizi nei confronti delle persone e quindi sostanzialmente ad andare in questa direzione.

per voi non valgono i lavoratori dipendenti e i pensionati, che devono continuare a pagare; voi siete i difensori degli evasori, di quelli che eludono il fisco e delle grandi compagnie che possono guadagnare e fare extraprofitti. Per questa ragione, voteremo contro il

Signor Presidente, signor Vice Ministro, colleghi, tredici mesi fa, il 22 giugno 2022, la Camera aveva già concluso l'esame di legge delega di riforma del fisco; certo, era il disegno di legge delega di un altro Esecutivo, di un Governo di unità nazionale, ma era anche il frutto di un'alleanza trasversale fra forze politiche diverse e spesso distanti, che però avevano trovato un punto di vista in comune su molti principi. Sappiamo come sono andate le cose: le forze politiche che poi sono risultate vincitrici alle elezioni hanno impedito che l'*iter* parlamentare si concludesse; nonostante ciò, larga parte di quel disegno di legge è stata traslata all'interno di questo disegno di legge di delega. Il primo dato che mi sento di osservare è che il Paese ha perso un anno di tempo per ragioni di puro tornaconto politico. Quel disegno di legge di delega poteva completare il suo *iter* sotto questo Governo, ma in questo caso avremmo i decreti attuativi e discuteremmo di questo, anziché tornare al tema della legge delega. Questo non è stato tanto un danno per l'opposizione, ma per il Paese, per le imprese e per le famiglie. Nonostante tutto quello che è accaduto, noi proviamo ad avere una logica oggettiva e a non utilizzare la lente dell'ideologia, quindi quello che è accaduto non ci impedisce di guardare con obiettività ai contenuti del provvedimento che siamo chiamati a votare. Certo, è strano che da parte di una forza di opposizione ci sia questa capacità di andare oltre le ideologie, di non dire un no preconcetto ed entrare nel merito, ma questo è il nostro modo di interpretare il ruolo di opposizione. Noi continuiamo a pensare che semplificare il fisco sia una necessità e un'urgenza *(Applausi)* e che questo sia il modo più efficace per combattere l'evasione. Forse è l'unico perché tutti i proclami nella lotta all'evasione hanno prodotto un nulla di fatto. La necessità di riformare il fisco è quindi un fatto ineludibile, che vogliamo condividere anche dai banchi dell'opposizione. Sappiamo però che il Governo è chiamato a un banco di prova importante, che non è quello di oggi, quello cioè di approvare una legge delega, ma è quello di fare in modo che i principi contenuti al suo interno producano risultati.

di superare gradualmente l'IRAP, di riformare la tassazione dei redditi finanziari, di razionalizzare le aliquote IVA, avvicinando i bilanci civilistico e fiscale, cosa che purtroppo ad oggi non è ancora avvenuta, e di dare anche finalmente concretezza ai principi dello statuto del contribuente, che credo sia la legge più calpestata della storia *(Applausi)*, perché sono anni che è entrata in vigore, ma è rimasta lettera morta. Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope abbiamo fortemente voluto la concretizzazione dello statuto del contribuente e il rispetto di quei principi e ci siamo battuti anche per la loro costituzionalizzazione, perché riteniamo che quella sia forse l'unica strada per fare in modo che quei principi diventino realtà e quindi si ricostruisca un rapporto di fiducia tra lo Stato e il cittadino, tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate. Questo però ancora non è accaduto: evidentemente. la maggioranza ha altre priorità. Devo però riconoscere al vice ministro Leo e al Governo nel suo complesso che un fatto apprezzabile è avvenuto: per una volta, non siamo di fronte ad un monocameralismo di fatto. C'è stata un'apertura significativa alle modifiche parlamentari parlamentari nelle Commissioni, alla Camera dei deputati prima, ma anche, parzialmente, al Senato. Questo credo sia un fatto positivo, perché vuol dire che non c'è solo un monocameralismo di fatto e non ci sono solo le questioni di fiducia sui decreti blindati, un altro mondo è possibile. Tenere in considerazione questo, nel prosieguo dell'attività di Governo, credo faccia bene alla politica e al ruolo del Parlamento e possa far bene anche al Governo.

dalle agevolazioni per i giovani alla detassazione dei premi di produttività, dalla riduzione dell'Ires per gli utili che vengono destinati a forme di partecipazione agli utili stessi da parte dei dipendenti, alla mensilizzazione del pagamento delle imposte per gli autonomi, alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative ai tavoli che saranno istituiti per l'emanazione dei decreti delegati. Credo che queste misure siano significative. Qui al Senato ci siamo battuti per un'altra misura alla quale teniamo molto: il principio secondo il quale, se si è assolti con sentenze irrevocabili perché il fatto non sussiste nel processo penale, questo deve fare stato anche nel processo tributario. *(Applausi)*. È una norma di civiltà che, insieme alle maggiori tutele previste per il contribuente nella fase del contenzioso, ci consegna un'amministrazione fiscale non più nemica dei cittadini e delle imprese. quindi a precisare che il nostro voto favorevole nasce da questa coerenza e dal fatto che i principi di delega sono sostanzialmente quelli individuati dal Governo Draghi. Apprezziamo l'apertura del Governo rispetto alle modifiche che abbiamo introdotto con il lavoro di Commissione. però a precisare che il nostro voto positivo, signor vice Ministro, non è una cambiale in bianco. La legge delega disegna una cornice, ma adesso starà al Governo riempirla e non è un'impresa di poco conto. Non siamo particolarmente ottimisti, perché la coperta è corta e i nodi arriveranno al pettine. C'è un problema di risorse, un problema che comincerà a manifestarsi già con la prossima legge di bilancio e non tutto si potrà magicamente risolvere. Noi vogliamo credere che su queste su queste tematiche, piuttosto che inseguire bandierine elettorali, proverete ad essere seri e coerenti con il mandato che vi ha dato il Parlamento. ancora una volta, l'opposizione abbia posizioni differenti. Noi preferiamo, alla ideologia, entrare nel merito e dare un'apertura di credito su una delega che avevamo costruito, avevamo concorso a definire. Spero che il Governo, nell'attuazione della delega, non ci faccia pentire di questo voto. Sarebbe un torto non a noi, ma al Paese. Vice ministro Leo, noi davvero attendiamo il Governo alla prova dei fatti, all'attuazione della delega. Non raccontiamo al Paese che con questa legge delega abbiamo ridotto le tasse, perché non è ancora avvenuto. Oggi, però, grazie a questa delega voi siete delle condizioni di poterlo fare. Fate dunque sentire la vostra voce attraverso i provvedimenti e non solo gli *slogan*.

non giriamoci intorno: questa legge delega non abbasserà le tasse per i cittadini e per le imprese di mezzo euro. Del resto, lo dimostrano i tanti diversivi che avete utilizzato durante questi giorni e nelle ultime settimane di discussione. quello che abbiamo ascoltato dal ministro Salvini, propone un condono delle cartelle esattoriali fino a 30.000 euro: un fuoco d'artificio, l'ennesimo, come sempre, per nascondere una delega che tutto ha in mente, fuorché alleviare le condizioni di lavoratori e imprese. Del resto, in questa direzione vanno interpretati anche i vagoni che avete aggiunto in corso d'opera a questa sgangherata locomotiva fiscale: la depenalizzazione della dichiarazione infedele per chi opta per l'adempimento collaborativo con l'amministrazione finanziaria, anche in presenza di comportamenti dolosi; l'estensione dello stesso adempimento collaborativo alle persone fisiche che hanno redditi oltre il milione di euro, anche se non stabiliscono la residenza in Italia, ma si limitano ad agire nel nostro Paese per interposta persona o attraverso un *trust*. Non c'è che dire, colleghi: è proprio la situazione in cui versa la maggior parte dei contribuenti italiani, preoccupati di far gestire le loro risorse che superano il milione di euro da un *trust*. Andate a raccontarlo alle 170.000 famiglie che avete liquidato con un SMS, cancellando il reddito di cittadinanza. Andate a raccontare loro che, mentre cancellavate l'unica forma di sostegno e di sostentamento che avevano, voi stavate approvando emendamenti per tutelare chi, comodamente dall'estero, fa gestire milioni di euro a un *trust*. Per ironia della sorte, *trust* vuol dire fiducia, quella stessa fiducia che voi state tradendo senza troppi ripensamenti. Io mi chiedo come pensiate di recuperare i 100 miliardi di evasione fiscale, se continuate a far passare il messaggio che le tasse siano pizzo di Stato. Questa delega Questa delega non abbassa le tasse di mezzo euro, perché non ha risorse a disposizione; perché, ancora una volta, questo Governo dimostra di non avere il coraggio di prendere le risorse lì dove ci sono. lì dove ci sono. Se la riforma fiscale deve avvenire ad invarianza di gettito, è chiaro anche a un bambino che, per abbassare le tasse ai lavoratori, al ceto medio, alle famiglie ed alle imprese, servono risorse. E l'Esecutivo cosa fa? Non trova niente di meglio che riproporre il taglio delle spese fiscali: sempre la solita chimera della storia fiscale italiana. Peraltro, lo stesso Governo, rendendosi conto dell'ennesima sparata, dice che, ovviamente, non si possono tagliare tutte le spese fiscali. Quindi, non si tagliano le spese fiscali fondamentali come le detrazioni sanitarie, le detrazioni per l'istruzione dei figli, per gli interessi passivi sulle rate dei mutui. Quindi, sul piatto resta davvero ben poco. ascoltato dire da un collega di maggioranza che nessuno ha criticato questa delega fiscale: davvero resto sbalordita ogni volta che provate a manipolare la realtà in questo modo. «Eravate presenti nelle Commissioni in cui si tenevano le audizioni?». Noi sì e in quelle audizioni abbiamo sentito le tante perplessità da Banca d'Italia, dall'Ufficio parlamentare di bilancio, dalla Corte dei conti. C'è stato anche un appello di fiscalisti guidati dall'ex presidente della Corte costituzionale Franco Gallo, che hanno espresso perplessità contro questa delega fiscale. Come si fa a dire che non ci sono perplessità? In realtà in questa delega vengono fuori nuovamente la pavidità dell'Esecutivo e la vostra subalternità alle *lobby*. Noi abbiamo fatto una controproposta, che abbiamo depositato come proposta alternativa, perché eravamo già certi che dei nostri emendamenti non ne sarebbe stato accolto nemmeno uno. Nella nostra proposta di delega fiscale abbiamo suggerito di abbassare le tasse ai ceti medi e bassi, ai pensionati, alle piccole imprese, e di recuperare risorse lì dove si sono generate enormi ricchezze e disuguaglianze, prima durante la pandemia, poi con la guerra. Abbiamo proposto di andare a tassare quindi gli extraprofitti, l'economia digitale e le transazioni finanziarie ad alta frequenza, tutte cose che voi non avete il coraggio di fare. come possa essere definita moderna una delega fiscale che, per esempio, non fa alcun cenno all'economia digitale. Voi state utilizzando gli stessi strumenti arrugginiti di venti anni fa: il concordato preventivo biennale e la *flat tax* erano già presenti nella proposta di delega fiscale dell'ex ministro Tremonti vent'anni fa, nei primi anni 2000.

pochissime imprese. Sono vent'anni quindi che proponete le stesse identiche ricette senza mettere la testa fuori da questo palazzo e rendervi conto che fuori c'è un mondo che drammaticamente è cambiato. Eppure, provate a presentare tutto come una svolta epocale con toni trionfalistici, come quando stappavate le bottiglie di *champagne* di fronte alla previsione di una crescita del PIL al 2023 del +1 per cento, senza poi ammettere che lo stesso Fondo monetario ha certificato un rallentamento e un crollo del ritmo di crescita del PIL: due giorni fa, infatti, vi è arrivata la doccia fredda con il PIL che, nel secondo trimestre del 2023, è in discesa. Non serviva del resto la sfera di cristallo per capire che un Governo dell'austerità, che punta solo ai tagli, sta dilapidando tutta l'eredità di crescita che noi vi abbiamo lasciato nel 2022 il Paese è cresciuto dell'11 per cento. Voi, però, avete tagliato tutti gli investimenti, avete tagliato il superbonus, Transizione 4.0 e ci avete riconsegnato alla stagnazione. Avete tagliato anche la spesa pubblica: davvero mi chiedo come possiate avere enfatizzato l'incremento di qualche miliardo del Fondo sanitario nazionale nella legge di bilancio,

prima della pandemia. È stata infatti pubblicata puntualmente nei giorni scorsi un'inchiesta sulla stampa che stima in 15 miliardi di euro nel 2024 la mancanza di risorse che andrà a gravare proprio sul Servizio sanitario nazionale a causa dell'inflazione. Passo brevemente all'inadeguatezza che avete dimostrato nella gestione del PNRR: ieri abbiamo ascoltato il ministro nella sua difesa lunare dei ritardi che ci sono sulla terza e la quarta rata. Ha detto che la Commissione europea ha accettato alcune modifiche, come se questo fosse un bollino di assoluzione per i ritardi e le incapacità che avete accumulato. Ancora una volta avete dimostrato che eravate sì pronti, ma solo ai proclami elettorali. Non ci rassicura nemmeno che i 16 miliardi di euro di progetti definanziati verranno recuperati nei fondi di coesione, perché lo stesso Ministro poi si è trovato costretto a dire che nulla è deciso, perché è ancora in corso una trattativa con l'Europa. E il Servizio studi della Camera ha pubblicato un *dossier* in cui si stigmatizza proprio l'assenza di risorse certe per finanziare questi progetti del PNRR. Colleghi, in conclusione, anche questa delega fiscale dimostra che il Governo non ha coraggio, non ha visione, non ha nulla sul piatto. Non ha alcuna ricetta per far crescere il Paese, perché sul piatto di questo Governo c'è solo un vuoto: c'è il baratro in cui state facendo precipitare il Paese.

più vicino ai contribuenti e alle imprese, più razionale e più amico. Grazie al disegno di legge delega che andremo ad approvare, il Governo, seguendo i principi contenuti nella delega, nei prossimi mesi avrà l'opportunità di cambiare radicalmente il rapporto tra fisco e cittadini ed eliminare l'odiosa percezione di un sistema fiscale troppo opprimente, a volte irrazionale o addirittura punitivo. Il lavoro che è stato fatto - di cui ringrazio il vice ministro Leo, il sottosegretario Freni, il presidente Garavaglia e la Commissione tutta - è stato molto puntuale puntuale e ha prodotto un testo che va nella direzione giusta. Dopo troppi anni servivano semplificazione e razionalizzazione. Al di là degli *slogan* e delle frasi fatte che ho sentito prima, ci sono misure concrete che verranno attuate tramite questa delega che i cittadini e le imprese aspettano da decenni. Grazie a questa delega ci sarà una razionalizzazione delle aliquote Irpef - è bene chiarirlo - e ci stiamo avvicinando a quello che è il nostro modello di *flat tax*: le quattro aliquote verranno diminuite possibilmente a tre, poi a due e così via. Quindi, si tratta di un percorso di razionalizzazione che porterà anche a una diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

che potrà essere rateizzato. Forse, per la prima volta in questo Paese, si pagheranno le tasse ad anno concluso e a reddito percepito e non su acconti e redditi che devono ancora essere incassati. Si passerà gradualmente a un'abolizione di quelli che erano gli studi di settore, che qualcuno aveva detto di aver abolito, ma di cui aveva solo cambiato nome chiamandoli ISA (Indici sintetici di affidabilità). Tramite questa delega si arriverà al graduale superamento anche degli ISA. Ci sarà anche l'abolizione dell'IRAP, tassa assolutamente odiosa e irrazionale che veniva pagata anche da chi non aveva redditi e da chi era in perdita. Solo, quindi, tutte misure concrete che verranno attuate nei prossimi mesi grazie all'approvazione di questa delega. Servirà poi anche il superamento della ritenuta d'acconto, che oggi viene pagata al 20 per cento: ci sarà la possibilità che questa venga ridotta e via via anche annullata. Ci sarà una rimodulazione delle aliquote IVA, più razionale a seconda delle tipologie dei beni di consumo. Ci sarà uno sfoltimento della giungla dei *bonus* e delle deduzioni (un difetto tipicamente italiano). Verrà poi introdotta una *flat tax* per le tredicesime e gli straordinari. Sono tutte misure concrete che vanno nella direzione di semplificare e ridurre il carico fiscale ai cittadini e alle imprese. proposito di imprese, parliamo anche di Ires: ci sarà la possibilità di introdurre maggiori detrazioni per i beni strumentali e maggiori detrazioni per le assunzioni, in maniera tale che di fatto l'aliquota Ires sarà inferiore al 24 che oggi le imprese pagano. Un altro dato che mi piace sottolineare: a differenza della bozza di delega che era stata affrontata con il precedente Governo,

questa delega getta i presupposti per diminuire le tasse e non per aumentarle. Oltre a una diminuzione di un carico fiscale che è effettivamente eccessivo, ci saranno anche una razionalizzazione e una semplificazione degli adempimenti fiscali:

per i redditi che ha denunciato in maniera chiara e trasparente. Oggi ci troviamo pertanto di fronte all'approvazione di un testo che è assolutamente positivo. Era una promessa elettorale del Governo e di tutto il centrodestra. Il Governo ci ha lavorato

dal Senato. Nei prossimi mesi ci troveremo di fronte a una serie di decreti attuativi che andranno nella direzione delle misure che ho appena citato e che sicuramente produrranno un nuovo rapporto tra il fisco e i cittadini, tra il fisco e l'impresa; un nuovo rapporto che non si baserà più su una sensazione di prevaricazione o comunque sulla percezione

grazie a questa delega finalmente - ripeto, dopo troppi anni - assisteremo a un cambiamento che definirei epocale e che va nella direzione giusta. *(Applausi)*. Signor Presidente, oggi discutiamo di una legge che conferisce al Governo un perimetro particolarmente ampio di intervento sulla materia fiscale.

Prima di entrare nel merito, penso che un'analisi onesta del sistema tributario non possa che partire da tre elementi. Il primo: le enormi sacche di evasione ed elusione fiscale, quelle che sottraggono alla collettività 100 miliardi l'anno, sono ben fotografate dal fatto che l'85 per cento dell'IRPEF proviene ed è esclusivamente sulle spalle dei pensionati e dei lavoratori dipendenti. elemento è la mancanza di equità orizzontale del nostro sistema di tassazione, per cui sul lavoratore dipendente pesa un dovere contributivo che è 1,6 volte più alto di quello di un percettore di dividendi; due volte superiore rispetto a chi dà in affitto i propri immobili con cedolare secca; 2,8 volte maggiore di quello di un professionista in regime forfettario. A complicare il quadro vi è il ginepraio di 626 diverse forme di detrazioni e deduzioni che incidono sui bilanci dello Stato per 125 miliardi l'anno: misure che è bene ricordarlo - solo in 19 casi producono sconti superiori al miliardo di euro e che in più della metà dei casi interessano non più di 30.000 contribuenti, prefigurandosi quindi come veri e propri abiti sartoriali per microcategorie. La questione della mancata equità orizzontale è stata acuita quest'anno dall'estensione della *flat tax.* A parità di reddito, un lavoratore dipendente versa al fisco 8.000 euro in più di un lavoratore autonomo che aderisce a questo regime fiscale. Fortunatamente, sul discorso della *flat tax* incrementale che presentava degli enormi problemi in termini di gettito fiscale, avete parzialmente corretto la rotta. Il terzo elemento è una pressione fiscale ancora troppo alta sul lavoro per redditi medio-bassi per coloro i quali provano a fare innovazione e, quindi, provano ad aumentare la competitività del nostro sistema produttivo. A nostro avviso, erano questi gli elementi sui quali bisognava lavorare: un radicale riordino delle detrazioni e un nuovo slancio nella lotta all'evasione; il tutto con l'obiettivo di restituire al fisco e quindi ai cittadini elementi di equità e È in questo segno che il Partito Democratico ha formulato le proposte: una revisione organica dell'Irpef nel segno della progressività, con un sistema ad aliquota continua come in Germania; facoltà diversamente mensili al posto dell'acconto e saldo per i soggetti ISA e precompilata per imprese e autonomi al posto di un concordato preventivo, su cui dirò meglio dopo; e ancora: la sostituzione della mini-Ires, con rafforzamento e stabilizzazione degli incentivi esistenti a partire dalla super ACE e dal superammortamento; incentivi per il reinserimento in Italia di attività produttive localizzate all'estero; il mantenimento dell'IVA ridotta per l'acquisto della prima casa e per gli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio esistente. Sono tutte proposte volte a rendere il fisco più vicino ai cittadini che pagano, a quelli che hanno difficoltà a pagare, ma sempre partendo dal presupposto che i comportamenti e le pratiche fraudolente non sono in alcun modo tollerabili. la strada che il Governo ha intrapreso va in tutt'altra direzione. Il Parlamento ha discusso questo provvedimento mentre all'opinione pubblica, nel pieno delle scadenze fiscali, si offrivano messaggi messaggi pericolosi e ambigui, come quello sulle tasse come pizzo di Stato, sulla necessità di porre fine a tutti i contenziosi sotto i 30.000 euro. Su questa premessa ideologica la strada scelta dall'Esecutivo non segue un disegno organico, ma tratteggia un quadro a macchia di leopardo, che antepone una logica corporativa al bisogno di equità, che dissemina il percorso di una serie di scappatoie per eludere il fisco. Si introducono norme che alterano la dinamica tra fisco e contribuenti, offrendo agli evasori e agli elusori la possibilità di giocare con l'erario, sanando le proprie posizioni un attimo prima che il fisco se ne accorga. Ci troviamo così davanti a un condono preventivo, a un auto-condono permanente; un primitivismo fiscale - come l'ha chiamato Rino Formica - in cui si rinuncia all'opportunità tecnologica per individuare con certezza la posizione fiscale di ogni contribuente e si opta per la contrattazione con l'imposta da pagare fissata per mezzo di un negoziato tra l'erario e il contribuente. Tutto questo avviene dopo che in meno di un anno si è data vita a dodici sanatorie, alcune anche particolarmente fantasiose, come quella sulle criptovalute, e altre particolarmente odiose, come la depenalizzazione di omesso versamento di IVA superiore a 250.000 euro. Non dimentichiamo l'aumento del tetto del contante, del tentativo di cancellare le sanzioni sui POS, dell'ordine del giorno portato da Fratelli d'Italia in Commissione sull'inappellabilità delle sentenze di primo grado sfavorevoli all'Agenzia delle entrate, per cento delle sentenze passate in giudicato vede lo Stato vincere e recuperare milioni di euro sottratti alla collettività. Oltre a questo, però, l'altro punto è l'anima corporativa di una riforma che sclerotizza e cristallizza l'idea di un regime fiscale diverso per ogni categoria di reddito: la *flat tax* per gli autonomi; un'imposta progressiva per i dipendenti e pensionati; un'imposta specifica per i possessori degli immobili; un'altra per i redditi finanziari; un sistema di concordato fiscale con predeterminazione dell'imposta per le piccole e medie imprese; un'imposta soggetta ad agevolazioni per società ed enti sottoposti all'IRES. È una scelta frutto di una frutto di una visione elettoralistica del Paese che lo incentiva a organizzarsi in corporazione al fine di ottenere ascolto ai propri interessi; il tutto a discapito dell'interesse generale che richiede, invece, una visione unitaria e il superamento di logiche particolaristiche. Paradigmatica in questo senso è la bocciatura della nostra proposta, a prima firma del nostro capogruppo Francesco Boccia, di inserire un fondo di perequazione nell'accordo di riordino dei tributi regionali che garantisse i LEP, con il divieto di finanziare i servizi alle persone, con l'aumento di tributi regionali fino al superamento della soglia della media della pressione fiscale nazionale. Il senso della nostra proposta era chiaro: in relazione all'autonomia differenziata i LEP si finanziano con la finanza centrale e comunque con il fondo di perequazione e non con nuove imposte regionali; un principio di assoluto buon senso su cui si è consumato uno scontro tutto interno alla maggioranza, dove alla fine ha vinto la Lega, dimostrando ancora una volta il vero scopo dell'autonomia differenziata. Si potrebbe continuare ancora, Presidente, ma io credo che il dato politico, il pericolo di questa riforma sia proprio qui: il fisco non come l'infrastruttura su cui far viaggiare il diritto alla salute, all'istruzione, ai servizi pubblici, ma come un'entità cattiva da guardare in cagnesco; l'evasione non come una forma di sottrazione ai propri doveri, ma come un atto di legittima difesa. La coesione sociale è come un inutile ostacolo rispetto al massimo beneficio individuale. avviene mentre si chiude la porta in faccia a 3 milioni di lavoratori poveri che attendono il salario minimo. Si notifica con un SMS a 169.000 nuclei familiari la revoca del reddito di cittadinanza. Si definanziano i progetti del PNRR che più impattano proprio sulle periferie e sul disagio sociale. Si tratta di un manifesto politico che perlomeno, Presidente, ha il dono della chiarezza: contro i poveri, gli onesti e soprattutto contro il Mezzogiorno, dalla parte dei furbetti e di un'idea regressiva dello Stato, non più chiamato a combattere, ma a certificare e semmai a favorire le diseguaglianze sociali e territoriali. Tutto questo merita la nostra più convinta opposizione.

questa mattina. Il Vice Ministro ha parlato tanto in queste settimane, anche attraverso i media e nelle Commissioni, agli italiani. E mi pare di capire, al di là della tecnicalità, che ci sono diverse riforme che il Governo sta provando ad intestarsi in questo mondo nuovo, in questo momento nuovo, dove nonostante tutto l'Italia sta andando molto bene. Abbiamo discusso del solco di questa riforma complessiva con i

nella storia della Repubblica lo sono stati con competenza rispetto a quello che il tema dell'interesse nazionale e della nostra coesione sociale, civile, economica e anche politica. Sugli appunti presi al volo,

hanno dato un contributo di idee e anche di preoccupazione. Gli aspetti fondamentali di questa riforma sono tre. Innanzitutto

a questa riforma che complessivamente riguarderà il contenzioso, quindi l'accertamento e tutto quello che ha spiegato bene, l'opera di *compliance* e soprattutto il concordato preventivo biennale. Tutto ciò restituisce il senso di una

aliquote nuove che accompagneranno il futuro economico di questo Paese. Pensiamo quindi a un sistema fiscale semplice, veloce ed equo. I costi della riforma nella prima fase riguardano accertamento, contenzioso a riscossione

non può essere più essere rinviata, collega Boccia - mi rivolgo direttamente a lei, non per il tramite della Presidenza - e che si inserisce anch'essa in una Siamo alla vigilia della ridefinizione del patto di stabilità in Europa, che non è non è secondario,

non regge rispetto alle complessità. I dati ci dicono che quest'anno pagheremo circa 100 miliardi di euro sul debito pubblico, il 50 per cento in più rispetto al 2022. Immaginiamo che, attraverso un fisco equo, più vicino e amico, una quota parte possa essere recuperata da una maggiore funzionalità dello Stato.

formule e ambizioni, con le tre nuove aliquote e tutto quello che in questa riforma è stato trattato e discusso. pensando a chi ci guarda da casa, spiegando agli italiani che uno Stato si regge insieme e, quindi, anche con il contributo di chi ha una *Weltanschauung* diversa dalla nostra.

cittadini e famiglie nel momento in cui lo Stato riuscirà a restituire, con una nuova organizzazione, velocità e modernità e quando i nostri figli, con uno Stato che recupera di più a livello tributario, potranno avere fiducia nel futuro. Guardiamo al Mezzogiorno: siamo in Parlamento e dobbiamo fare i deputati nazionali. Molto spesso si parla del Sud che viene descritto come "non ancora Nord", non conoscendolo. Vale quello che ha detto il ministro Fitto nei giorni scorsi, parlando del PNRR. Al Sud ci sono tante risorse dell'obiettivo convergenza, ma mancano le imprese,

Bisogna essere attrezzati a essere classe dirigente. Mi stupisce che oggi alcuni sindaci, che dovrebbero conoscere i provvedimenti dello Stato, si sveglino, avendo anche assessori alle politiche sociali, senza essere preparati a ricevere tutti tutti i fuoriusciti dal sistema del reddito di cittadinanza, che devono essere accolti e accompagnati, al di là della comunicazione dell'INPS. uno Stato più veloce, uno Stato più equo nella raccolta della tassazione e tutti contribuiremo meglio, immaginando che questo percorso è giusto, perché alle diverse latitudini avremo più investimenti; per cui la parte più interessante è anche attrarre quei capitali esteri che hanno guardato...

finanche in Africa, dove il piano Mattei, unito alla nuova tassazione italiana, rappresenta la nuova frontiera di un'Italia, che noi che veniamo dal Sud proviamo a guardare in positivo, rovesciata. Quindi, grazie del buon lavoro, vice ministro Leo. Il contributo penso sia positivo e in dichiarazione di voto i colleghi esprimeranno il voto

Signor Presidente, desidero innanzitutto rivolgere un sincero ringraziamento a tutti i rappresentanti delle forze parlamentari presenti in quest'Aula. Il lavoro che è stato fatto non è di una parte politica, seppure una parte politica abbia creato la struttura portante di questo provvedimento, ma c'è stata condivisione su tanti punti con le forze di opposizione.

quando un provvedimento analogo fu messo a terra da studiosi del calibro di Bruno Visentini, di Cesare Cosciani, di Gino De Gennaro. Fu un provvedimento che segnò una svolta, nel passaggio da una economia di tipo agricola ad un'economia di tipo industriale. E questo lo si fece lo si fece grazie soprattutto a un intervento in materia fiscale che ridisegnò i tributi. Come ricorderete, fu introdotta l'IVA in luogo dell'IGE e furono introdotti tributi personali in luogo dei tributi reali. Noi abbiamo tentato di fare la stessa operazione, che abbiamo strutturato in quattro parti, perché non vogliamo neanche essere tacciati come quelli che vogliono creare problemi alla finanza pubblica. Abbiamo organizzato questa delega fiscale in quattro aree. Una prima area che riguarda i principi, quelli di diritto interno e quelli di diritto internazionale.

un aspetto fondamentale, cioè che servono i tempi tecnici per fare ciò: i passaggi parlamentari ed un eventuale *referendum*. Quindi, abbiamo fatto in modo di dire che in questa delega lo statuto del contribuente deve rappresentare una sorta di pre-legge a tutto il sistema tributario

soprattutto al legittimo affidamento del contribuente, alla certezza del diritto e alla semplificazione. Proprio sulla certezza del diritto noi abbiamo speso tanti interventi. Se voi leggete, come avrete fatto, il testo della delega, vedrete che abbiamo posto l'accento sul rendere molto più confidente il sistema tributario per i contribuenti, per gli addetti ai lavori e per la stessa amministrazione finanziaria.

È possibile immaginare che questo sistema sia molto attrattivo per gli investitori esteri? È stato detto che qui si vogliono favorire i soggetti che vengono dall'estero

Questo è l'obiettivo che si intende perseguire con questa delega. La semplificazione. La collega Mennuni ha prima puntualmente ricordato la Babele di istruzioni al modello di dichiarazione dei redditi: oltre mille pagine. È possibile riuscire a districarsi in questo magma assolutamente ingestibile della materia tributaria? Ecco perché noi dobbiamo intervenire. Lo dobbiamo fare nell'interesse del Paese, nell'interesse dei cittadini, nell'interesse di tutti.

quello che è il reddito che risulta dai dati di economia nazionale e il reddito dichiarato) che oscilla tra i 75 e i 100 miliardi di euro. Si può dire, quindi, che è stata fatta lotta all'evasione nel corso del tempo, dal 1990 al al 2021, perché nel 2022 dobbiamo dare atto all'Agenzia delle entrate che è stato fatto un recupero importante anche se, nonostante ciò, abbiamo sempre questo differenziale. Come si deve intervenire, se non cambiando rotta sull'accertamento?

Chi vi parla era al Ministero delle finanze, quando c'era il ministro Formica: da allora ad oggi è passato tanto di quel tempo che oggi abbiamo la tecnologia, abbiamo l'informatica. Abbiamo circa 2,2 miliardi di fatturazioni elettroniche; abbiamo abbiamo le dichiarazioni precompilate; abbiamo l'intelligenza artificiale e l'analisi predittiva. Siamo in grado di dire millimetricamente al contribuente Maurizio Leo: «Questo è il suo reddito e, e, fermi restando gli adempimenti IVA, se lo dichiari e quindi accetti la proposta che ti fa l'amministrazione finanziaria, per due anni starai tranquillo». Questo è il cambio di rotta nella lotta all'evasione, questo è il modo di contrastare i famosi 75-100 miliardi che rappresentano un fardello per la nostra economia.

l'enorme ammontare di evasione fiscale. Diversamente, potremmo stare per anni a discutere di lotta all'evasione, come si è fatto dagli anni Novanta a oggi, ma non si abbatterà mai questo importante carico che abbiamo.

Se leggiamo bene i testi normativi, per quanto riguarda la parte del reddito da lavoro dipendente diciamo che vogliamo mettere assolutamente sullo stesso piano il dipendente e il lavoratore autonomo. Come lo facciamo?

è necessario trovare e reperire le risorse. Vogliamo dire che, se il dipendente ha certe spese che sono obiettivamente sostenute (penso alle spese per la mobilità, la mobilità, per la formazione), queste devono essere dedotte integralmente nella determinazione del reddito da lavoro dipendente. Abbiamo detto che, se vengono fatte delle erogazioni liberali da parte del datore di lavoro al lavoratore dipendente - già lo abbiamo fatto nella legge di bilancio - possiamo elevare il tetto a quindi maggiori risorse in mano ai lavoratori dipendenti. Lo stesso abbiamo fatto per la tredicesima mensilità: se la tredicesima mensilità, soprattutto per le fasce più deboli, viene assoggettata a una tassazione più mite quindi non a una tassazione progressiva, consentirà un potenziamento dei consumi. Ovviamente il soggetto che ha redditi da lavoro dipendente più bassi non terrà in tasca le risorse che ha risparmiato con la fiscalità, ma sicuramente le userà per comprare regali per i figli, per la famiglia e via dicendo. Quindi, le immetterà in un circuito virtuoso. Infatti il soggetto che venderà questi beni pagherà IVA e pagherà imposte sui redditi. Ecco come pensiamo di cambiare anche il reddito di lavoro dipendente, per gli straordinari che eccedono una certa soglia e per i premi di produttività. Non ci si può tacciare di guardare con favore ad un'area della nostra economia e di non guardare con altrettanto favorevole al mondo del lavoro dipendente. Vi un altro tema che mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione, che è quello della riscossione. Oggi abbiamo - l'ha ricordato il direttore dell'Agenzia delle entrate - 1.153 miliardi di carico presso l'Agenzia delle entrate-riscossione e questo carico si alimenterà sempre di più. Se non mettiamo mano a questo a questo settore, non riusciamo a venirne fuori. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dire che se viene affidato il carico dall'ente impositore all'Agenzia delle entrate-riscossione e nei cinque anni successivi, nonostante gli sforzi fatti dall'Agenzia delle entrate, queste somme non si riscuotono, allora le si devono restituire all'ente impositore, perché si tratta di soggetti falliti, deceduti e via dicendo. Non si può lasciare in piedi questa situazione che è Ecco come vogliamo orientarci: vogliamo rivedere il sistema del contenzioso. Questo ce lo dice l'Europa; ci stiamo muovendo nella logica di seguire quello che ci viene detto dall'OCSE, dal Fondo monetario internazionale e dall'Europa. L'altro tema riguarda il contenzioso tributario, su cui sto insistendo e ringrazio tutti voi che avete avuto la sensibilità di capire l'urgenza di questo provvedimento, perché uno dei tasselli fondamentali del PNRR è rappresentato dalla riforma del contenzioso. Nella passata legislatura si è fatto abbastanza con la legge n. 130 del 2022, ma l'Europa ci dice che dobbiamo spingere di più e accelerare sulla riduzione del carico del contenzioso. Tutti questi elementi noi li abbiamo inseriti tra i criteri direttivi della delega.

proposta che guarda con particolare interesse alle Regioni a statuto speciale. Noi non possiamo accoglierlo, ma saremo sicuramente favorevoli a valutare la possibilità, nella prossima legge di bilancio, di inserire delle indicazioni in questi termini. Chiudo ringraziando ancora una volta tutti i rappresentanti delle forze parlamentari e penso che tutti insieme stiamo scrivendo una pagina veramente importante nella storia economica di questo Paese.

noi ravvisiamo un rischio di sostenibilità sociale nel momento in cui il Governo svuota con una serie di provvedimenti l'impatto l'impatto dell'Irpef sulle entrate dello Stato e trasferisce competenze agli enti territoriali, andando così a definanziare le entrate complessive dello Stato. Con questo emendamento - lo ripeto - chiediamo di preservare la centralità fiscale dello Stato.

l'evasione fiscale e noi, con l'emendamento 2.16, più che ridurre l'evasione fiscale la vorremmo contrastare con qualunque strumento e con qualunque modalità e quindi chiediamo, nell'ambito di questa proposta, che il Governo sostituisca la parola «riduzione» con la parola «contrasto».

Presidente, con l'emendamento 2.20 chiediamo innanzitutto la diffusione dei pagamenti elettronici, anche perché è proprio di questi giorni la conclusione di un protocollo tra ABI e i servizi elettronici di pagamento. Chiediamo quindi, al fine di contrastare l'evasione fiscale, un maggiore ricorso ai pagamenti elettronici

Presidente, al fine di favorire lo sviluppo del terzo settore, con l'emendamento 2.26 proponiamo l'istituzione delle imprese cosiddette di comunità, anche per contrastare i fenomeni di spopolamento economico soprattutto nei piccoli centri urbani.

noi vorremmo un rafforzamento di tutta la digitalizzazione del sistema tributario. Vorrei ricordare che solo nel 2019, quando nel corso del Governo Conte II introducemmo, confermammo e prorogammo la fatturazione elettronica, molte forze di centrodestra erano addirittura contrarie

di evasione fiscale nell'anno 2021-2022. Quindi noi chiediamo un rafforzamento della digitalizzazione di tutto il sistema tributario.

altresì una maggiore detassazione dei redditi a favore di investimenti a tutela dell'ambiente, a sostegno delle produzioni di energia da fonti rinnovabili e degli impianti di autoconsumo dei processi produttivi di energia. sul tema con una serie di emendamenti che poi caratterizzano il seguito di questo articolo 2.

dando la possibilità allo stesso di verificare periodicamente le informazioni contenute nelle diverse banche dati dell'Agenzia delle entrate e degli uffici tributari. Nello stesso tempo vorremmo incoraggiare un uso migliore del contraddittorio tra Agenzia delle entrate

necessaria al contribuente per verificare anomalie o rischi di evasione fiscale, in modo tale da consentire un uso preventivo degli strumenti a disposizione dell'Agenzia,

Presidente, in merito all'emendamento 4.24, noi chiediamo, al fine di garantire ai contribuenti una migliore conoscibilità della giurisprudenza in materia di diritto tributario ed una maggiore prevedibilità

andando a ridurre ulteriormente gli scaglioni di reddito e quindi le aliquote fiscali da tre a due, ma anche per tutta una serie di micro imposte sostitutive proporzionali, non progressive, che introduce nella riforma fiscale. Nell'ambito di questo emendamento, noi esprimiamo la contrarietà a questa intenzione del Governo, oltre a chiedere quella di innalzare la soglia della *no tax area* dei redditi da lavoro dipendente fino a 12.000 euro.

di semplificazione delle aliquote che vanno verso la *flat tax*. Questo emendamento contiene il cuore della nostra proposta, che prevede invece un sistema di tassazione duale, per cui i redditi da lavoro vengono tassati secondo una Irpef progressiva continua sul modello tedesco, mentre gli altri redditi vanno verso altre forme di tassazione. Siamo altresì contrari, come già detto in discussione generale, alla proliferazione di cedolari e imposte sostitutive e questo emendamento ribadisce questo principio in delega.

non solo chiediamo la soppressione nella prospettiva dell'imposta unica, ma ravvisiamo che anche in questa prospettiva, che è irrealizzabile - così come peraltro già ribadito anche dalla Ragioneria generale dello Stato che ha

determini il rischio di mancanza di sostenibilità finanziaria per le entrate e per le coperture finanziarie. Inoltre, la stessa introduzione della *flat tax* minaccia anche la sostenibilità sociale,

dello Stato sociale, che peraltro il Governo ha già introdotto con diverse forme nella legge di bilancio e da ultimo proprio con il taglio dei percettori del reddito di cittadinanza occupabili, oltre ai tagli sugli investimenti (vedasi Transizione 4.0), nonché i tagli sulla sanità in rapporto al PIL e ad altre misure a sostegno dello Stato sociale. Noi intravediamo dunque un grande rischio la conservazione di quello Stato sociale che ha fatto grande l'Italia in tutti questi decenni.

all'evasione fiscale, dato che sulle spese sanitarie c'è molta evasione da recuperare che si nasconde.

all'estensione della cedolare secca sugli immobili strumentali *tout court.* Quindi gli emendamenti propongono una serie di correttivi volti a redistribuire questo vantaggio fiscale non solo a favore dei proprietari degli immobili, favorendo in questo modo

con l'emendamento 5.54 poniamo al Governo un problema, ovvero come adeguare i salari al mutato potere di acquisto della moneta e quindi al tema dell'inflazione. quest'ottica l'introduzione di meccanismi di adeguamento dei salari all'inflazione che oggi sta erodendo il potere di acquisto soprattutto dei lavoratori che non hanno la possibilità di avere

ricordiamo al Governo che esistono anche le imprese e che esistono anche strumenti fiscali incentivanti. Il tema è quello noto anche come superammortamento. Proponiamo la sostituzione del comma a) con una riformulazione e la conseguente soppressione del punto b). Ciò significa che suggeriamo che la legge delega dovrebbe prevedere strumenti incentivanti per gli incrementi netti sia del patrimonio, sia dell'occupazione che deriva da contratti a tempo indeterminato, nonché la stabilizzazione dei crediti di imposta con priorità alle piccole imprese, in particolare per gli investimenti qualificati nei nuovi beni strumentali e che riguardino i tre pilastri, cioè la transizione ecologica, l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo e la formazione, soprattutto soprattutto laddove riguardi il Mezzogiorno. Non comprendiamo le ragioni per le quali il Governo si dimentica delle imprese e non aderisca invece a questa formulazione che in qualche modo amplia la formulazione prevista nel testo A della legge.

di ridurre l'aliquota IRES a beneficio delle imprese che adottano sistemi di gestione certificati a favore dell'ambiente, andando a riconoscere un credito d'imposta in modo tale che l'agevolazione venga destinata alla realizzazione di impianti che producono energia da fonti rinnovabili, oltre a politiche attive del lavoro.

impegna il Governo, nelle more dell'adozione degli interventi di revisione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, a valutare l'opportunità di adottare i necessari atti volti ad un

di adottare i necessari atti volti ad aumentare le compensazioni dell'IVA applicabile agli animali, specie bovini e suini, in modo tale da consentire alle imprese di poter usufruire di queste agevolazioni e di poterle compensare.

Signora Presidente,attraverso l'ordine del giorno G7.300 noi segnaliamo una necessità importante. In un momento di grave difficoltà e di carenza di liquidità da parte delle aziende agricole, soprattutto di quelle zootecniche, che sono fondamentali,

il vice ministro Leo e il sottosegretario Freni, per la loro attenzione. L'ordine del giorno G7.300 è propedeutico ad un'azione congiunta, che spero non sia solo della maggioranza,

in merito all'imposizione fiscale delle autovetture e delle flotte aziendali. Da una parte, chiediamo l'introduzione di una tassa di immatricolazione parametrata al costo dei veicoli e sulle emissioni di CO2; dall'altra, chiediamo anche la revisione della deducibilità fiscale del costo delle autovetture aziendali, parametrate sempre all'emissione di CO2 e al chilometraggio percorso dai mezzi, in modo tale da facilitare e da favorire il chilometro zero.

di intervenire sul catasto, dando una riformulazione totale alla questione catastale. Se, infatti, si vuole affrontare il problema di equità dal punto di vista fiscale, vi è da affrontare anche il problema del valore degli immobili, visto che l'Italia è un Paese dove le proprietà immobiliari sono molto diffuse.

con l'emendamento 8.0.2, noi chiediamo uno spostamento della tassazione dai fattori della produzione, ovvero lavoro e imprese, su tre aspetti sui quali oggi si accumula la ricchezza, ovvero gli extraprofitti, l'economia digitale

per consentire la convocazione delle Commissioni, in particolare di quelle impegnate nell'esame dei decreti-legge in calendario, sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15,30.

Signor Presidente, i nostri emendamenti all'articolo 9 sono tutti volti a contrastare il proliferare delle imposte sostitutive, in particolare per gli effetti negativi che hanno sulle addizionali di Comuni e Regioni. Chiediamo le nostre proposte emendative che anche le imposte sostitutive possano contribuire al gettito degli enti locali che, come abbiamo visto, sono fortemente penalizzati dalla delega.

aggiungo la mia firma all'emendamento 13.301 che, al pari dell'emendamento 13.303, chiede che l'attivazione di un fondo per equativo in favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante, per garantire la copertura integrale dei LEP,

per chiedere che il livello dei tributi dei territori con meno capacità fiscale non superi il livello medio nazionale di tassazione, perché ci preoccupa il fatto che le Regioni con meno capacità fiscale dovranno alzare le tasse per garantire i servizi pubblici ed è inaccettabile che per gli stessi servizi

Tra l'altro, prendiamo atto con stupore che alcuni colleghi di Fratelli d'Italia prima in Commissione e questa mattina in Aula si dicevano favorevoli a questo emendamento, salvo poi accettare supinamente le decisioni della Lega. un'occasione di libertà e di dignità per senatori, affinché possiamo aiutare le Regioni e i territori che stanno più indietro e non spaccare l'Italia, come volete fare.

che si è limitato ad una difesa di parte dell'operato svolto, senza dare nessuna indicazione su misure concrete per sostenere le famiglie e le imprese dei numerosi territori che purtroppo hanno subito calamità naturali rilevanti: direi di parlare dell'intero Paese. L'emendamento, che è stato dichiarato inammissibile, e personalmente non ne comprendo le ragioni, le ragioni, è invece particolarmente rilevante, perché mira ad introdurre una proroga delle scadenze di diversi adempimenti fiscali che interessano il lavoro e l'impresa, spostandoli dal 31 luglio al 21 agosto. Su tale questione, anche pubblicamente, erano emersi grandi consensi da parte anche di forze politiche della maggioranza, che si erano da subito precipitate a garantire ai cittadini che ci sarebbe stata una proroga degli adempimenti fiscali. Invece, in quest'Aula, continuiamo ad assistere ad un silenzio incomprensibile, soprattutto perché vengono a mancare le risorse per dimostrare la vicinanza e l'attenzione dello Stato nei confronti delle famiglie e delle imprese colpite dalle calamità. Non ci accontentiamo del nulla. Con questo emendamento avremmo dimostrato che lo Stato è vicino ai cittadini e invece la maggioranza continua a lavorare in maniera molto distante dai problemi reali delle imprese, favorendo ponti per gli evasori e dimenticandosi del lavoro e dell'impresa. Così si rallentano gli investimenti pubblici e privati e si porta l'Italia in recessione. Porterete anche questa responsabilità insieme alla disattenzione che avete nei confronti dell'Italia che lavora e produce.

è una situazione veramente drammatica quella che sta vivendo la nostra Regione. Ieri il ministro Musumeci è venuto a parlare e penso che la linea politica del MoVimento 5 Stelle sia stata espressa in maniera forte. In questo provvedimento si sarebbero utilizzare ampi spazi per inserire il tema: chiedo al Governo di fare un'attenta riflessione prima di proseguire su questa linea. *(Applausi).*

Lo sappiamo benissimo, colleghi: avete fatto quest'emendamento perché volete fare un comunicato stampa dicendo che vi hanno bocciato la possibilità di trovare trovare le risorse *(Applausi).* E poi mi venite a dire anche che non è strumentale? Abbiate almeno il coraggio di far finta di niente! In una legge delega mettiamo la proroga di alcuni interventi di beneficio o meno? La Presidente del Consiglio dei ministri è stata chiara: gli interventi e le proroghe necessari saranno fatti con provvedimenti *ad hoc*, non certo in una legge delega.

focalizzato il suo intervento - com'era giusto che fosse - sulle popolazioni colpite dalle calamità, che sono tante e versano nelle condizioni che tutti conoscete.

tutte le associazioni di tributaristi italiani - di spostare per sempre quel termine al 21 agosto 2023, senza l'applicazione di sanzioni o interessi, e lo sapete. Lo sapete così bene che i giornali specializzati in Italia erano pieni di interviste a esponenti della maggioranza che garantivano che sarebbe avvenuto già durante la discussione in Commissione finanze. che l'emendamento sia stato ritirato. Noi lo dobbiamo ripresentato in Aula e faccio ancora fatica a capire perché sia inammissibile, perché qui stiamo parlando della definizione di una scadenza non solo per quest'anno, ma per sempre. Ovviamente il rappresentante del Governo ora ci spiegherà quali sono le ragioni per le quali non è intervenuto.

ringrazio per gli interventi, ma penso sia opportuno fare un po' di chiarezza sul tema. Abbiamo una situazione contingente in ordine alla quale siamo assolutamente d'accordo a rimettere in termini tutti i contribuenti e i professionisti che li assistono che non hanno potuto osservare gli adempimenti. A tale riguardo c'è stato un comunicato stampa del MEF nel quale è stato detto che la remissione in termini potrà essere fatta non appena avremo perimetrato bene l'ambito delle zone colpite dalle calamità. Questa è la situazione La situazione a regime quale sarà? Abbiamo un testo che rivede tutto il calendario degli adempimenti perché - come abbiamo detto - assistiamo oggi a una situazione un po' a macchia di leopardo, perché i versamenti possono essere fatti a una certa data, le dichiarazioni a novembre. Abbiamo detto di rivedere tutto il calendario degli adempimenti riportare le lancette indietro. Diciamo che la modulistica deve essere predisposta sessanta giorni prima rispetto al momento in cui bisognerà effettuare gli adempimenti; poi bisognerà fare la modulistica e in quel contesto ci faremo sicuramente carico delle situazioni cui si verificano eventi calamitosi. Questa è la situazione. Per la vicenda contingente c'è già un impegno del Governo nel dire che, non appena avremo il quadro di riferimento, rimetteremo in termini i soggetti che non hanno potuto osservare gli adempimenti. Per il futuro sicuramente ne terremo conto in sede di decreti legislativi. senatori Turco 14.0.300. Ricordo al Vice Ministro che il Governo non ha rinviato - così come è stato sempre fatto - le scadenze dei versamenti di luglio ad agosto senza sanzioni e senza interessi.

Presidente, questo articolo, che ha assorbito l'ex articolo 14, si dedica al tema della riscossione. Noi ci siamo pronunciati in Commissione più volte in maniera assolutamente contraria al superamento degli ISA. In particolare vorrei illustrare l'emendamento 16.306, in cui proponiamo per i soggetti che hanno indici sintetici di affidabilità fiscale il superamento del meccanismo di acconto e saldo con un versamento mensile, che dal nostro punto di vista agevolerebbe questo tipo di contribuenti premiandoli per l'affidabilità.

«delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari, che non possono in ogni caso eccedere complessivamente la misura della sorte capitale, degli interessi e di ogni relativo accessorio sino all'effettivo soddisfo,».

sull'emendamento 20.0.300, che prevede l'aggiunta di un articolo volto ad istituire un fondo perequativo in favore dei territori con maggiore capacità fiscale per abitante, per abitante, al fine di garantire il superamento di disuguaglianze che potrebbero mettere a rischio l'effettiva tutela dei livelli essenziali delle prestazioni nei territori svantaggiati. il Governo, o almeno un esponente della maggioranza, ci dicesse in che modo il Governo intende garantire in tutto il territorio nazionale, a tutti i cittadini, l'effettivo accesso ai livelli essenziali delle prestazioni di cui alla lettera *m)*, dell'articolo 117 Questa domanda non suoni come retorica, perché noi, mentre siamo in Aula a discutere della delega fiscale, siamo anche in Commissione impegnati a discutere un disegno di legge che vorrebbe anteporre l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, cioè l'autonomia differenziata, all'effettiva e piena realizzazione di quanto previsto dall'articolo 117, cioè la piena ed effettiva tutela dei livelli essenziali. Di fronte alle nostre ripetute critiche in ordine a questa inversione logica e anche di fronte alle perplessità che hanno sollevato giuristi come Giuliano Amato, Franco Bassanini, Franco Gallo e Pajno, noi non abbiamo ricevuto alcuna risposta. In questo caso capita che il Governo dia anche parere negativo ad un emendamento che vorrebbe dire che comunque bisogna reperire le risorse per far sì che in tutta Italia siano davvero garantiti questi livelli essenziali. Se questo emendamento non va bene e se il Governo, come ci sentiamo dire in Commissione, vuole garantire effettivamente l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, ci potreste dire in Aula dove pensate di reperire le risorse? In che modo pensate di dare attuazione all'articolo 119? In che modo voi garantite che prima si attuino i livelli essenziali e dopo, eventualmente, si proceda ad assicurare forme di autonomia differenziata?

di una riforma fiscale che vorrebbe ridurre la capacità di spesa dello Stato e l'attuazione di un'autonomia differenziata che antepone la differenziazione alla piena attuazione dei livelli essenziali rischia davvero di compromettere l'unità del Paese e l'effettivo esercizio di diritti fondamentalissimi.

Il tema dell'autonomia verrà opportunamente affrontato a tempo debito con i tempi e gli approfondimenti necessari. Oggi stiamo parlando di una delega fiscale che, tra l'altro, ha affrontato in maniera molto approfondita ciò che riguarda il finanziamento degli enti territoriali, approvando tantissimi emendamenti; avrete avuto modo di vederli anche nei documenti che arrivano da suggerimenti delle Regioni, dei Comuni, delle Province. Quindi si è fatto anche un grande lavoro su questo aspetto. Il tema dei LEP sappiamo che esiste da tempo, bisogna distinguere due piani. Il fatto che una differenziazione nel nostro Paese esiste e che storicamente non è stata affrontata non necessariamente impatta nell'immediato sulla finanza pubblica; pubblica; impatterà solo nel momento in cui verranno fatti i calcoli esatti. Ma questo non ha niente a che vedere con i meccanismi generali di finanziamento di Comuni, Province e Regioni, che sono stabiliti perfettamente dalla Costituzione. *(Applausi)*.

la risoluzione ad una serie di problematiche in tema di autonomia differenziata. Innanzitutto, in questa delega fiscale non c'è menzione del come andare a finanziare l'autonomia differenziata e i livelli essenziali delle prestazioni. non si va a determinare il fabbisogno finanziario. In tema di fondi di perequazione, non vengono definiti i criteri di determinazione né lo stanziamento di alcuna risorsa. infine irrisolti i temi relativi soprattutto ai residui attivi che potranno essere determinati a seguito dell'assegnazione di prestazioni alle Regioni. Per tutte queste ragioni chiediamo di sottoscrivere questo emendamento e lo sosteniamo.

Non ci sarà più il fisco che ti convoca, ma ci sarà un fisco che viene a casa tua. È un rapporto completamente diverso, collaborativo rispetto a quello che è stato fino ad oggi non tanto per i provvedimenti, quanto per la percezione

rappresenta un elemento fondamentale perché diventa principio generale e fondamentale del rapporto fisco-contribuente. La semplificazione è un elemento fondamentale importantissimo in modo tale da poter sfuggire a quella miriade e miriade di norme e cavilli che fino ad ora hanno inchiodato e rallentato non solo del contribuente, ma anche quella delle imprese e delle aziende che magari dall'estero volevano venire sul nostro territorio. La mancanza di certezza di quelle che fossero le regole e la miriade di provvedimenti presenti spaventavano gli investitori tanto da indurli a non venire in Italia.

la lotta all'evasione; va cambiata la lotta all'accertamento che quindi deve essere fatta in maniera completamente diversa. Partiamo da un presupposto: non tutti sono evasori. non tutti sono evasori. *(Applausi)*. Una persona che dichiara quali sono i balzelli che dovrebbe pagare e poi non riesce a farlo non è un evasore, ma una persona che non è riuscita a pagare. Un fisco che sia accanto al contribuente e che possa aiutarlo e sostenerlo nel pagare quello che giustamente deve pagare allo Stato è un fisco che ti sta accanto e che tu non vedi più come nemico. Il fatto di poter pagare le tasse distribuite su una annualità in maniera diversa, il fatto di non pagare più l'anticipazione e di poterlo fare in maniera rateale, partendo dal primo gennaio dell'anno successivo, sono tutti quanti provvedimenti che vanno in tal senso. Cosa accade

È stato fatto prima riferimento alle zone ZES. Abbiamo infatti una parte dell'Italia che può essere può essere trasformata e valorizzata in maniera assoluta e fondamentale; realizzare dei provvedimenti normativi che consentano defiscalizzazione per chi va a investire su quei territori significa creare su di essi ricchezza. La ricchezza da parte dello Stato, poi, qual è?

A cosa mirano i princìpi costituzionali di progressività del sistema tributario e di capacità contributiva? A me sembra chiaro il dovere di concorrere alle spese pubbliche richiamato negli articoli 2 e 3 della Costituzione secondo il principio di solidarietà e di uguaglianza di tutti i cittadini dello Stato italiano. La funzione principale del fisco è per noi il superamento delle disuguaglianze e la solidarietà sociale. Le disuguaglianze nel nostro Paese sono aumentate e, dopo la crisi energetica e pandemica, hanno aggravato l'ingiustizia sociale, che era già enorme. Secondo il rapporto Oxfam, la pandemia ha aumentato le disuguaglianze, mentre

La delega non interviene per riequilibrare questo squilibrio, non tocca le basi imponibili che in questo momento sono tassate in maniera diffusa e poco progressiva, anzi fa esattamente il contrario. Ma c'è di più: la valutazione della capacità contributiva dovrebbe essere considerata secondo la situazione complessiva del patrimonio del contribuente, invece non è così.

sempre di più nella possibilità di cambiare la propria condizione materiale di partenza. È evidente che in questo contesto un ruolo fondamentale sarebbe da assegnare alla lotta all'evasione fiscale.

dei quali 15 miliardi sono ascrivibili alle evasioni internazionali dei grandi gruppi, non si può sentir parlare di evasione di necessità. Non si può sentir parlare di quello che ho sentito prima, ovvero del fatto che bisogna essere vicini al contribuente che non è in condizioni di pagare.

nella legge di bilancio e si arriverebbe così a una sorta di condono preventivo, nonché ad un vero e proprio condono penale. Il risultato è un incentivo ad evadere. Questa impostazione è completamente sbagliata, a nostro avviso, e andrebbe totalmente ribaltata. La strada maestra deve essere quella di i controlli e punire gli evasori. L'unico meccanismo premiale deve essere rivolto ai contribuenti onesti, che assolvono il proprio dovere con il fisco, proprio come fanno i lavoratori dipendenti e i pensionati. Fatemelo dire: la *flat tax*

i lavoratori dipendenti e i pensionati continuano a pagare: paga Pantalone, come si usa dire. Occorrerebbe fare il contrario, introdurre invece un meccanismo, come abbiamo proposto nei nostri emendamenti, di progressività molto ravvicinata, quindi con degli scalini molto bassi, per favorire i redditi da pensione e da lavoro dipendente. Questo è il modo per dare un peso significativo anche alle retribuzioni e per favorire la retribuzione dei lavoratori e dei pensionati. Lo ripeto: il

In particolare, la difficoltà nel trovare lavoro c'è nel Mezzogiorno, ma si continua a pensare che quelle persone non abbiano voglia di lavorare. Questa è l'idea di molti di voi nella maggioranza: arrangiatevi e fate quello che volete! Lo Stato vi scarica: al massimo andate dai Comuni. Questa è l'idea che avevate trenta anni fa,

Signor Presidente, signore e signori del Governo, onorevoli colleghi, l'approvazione del disegno di legge di delega sulla riforma fiscale è il secondo tentativo il secondo tentativo in due anni di corrispondere agli impegni che l'Italia si è assunta in sede di approvazione del PNRR, posto che la riforma è stata indicata come di accompagnamento. Anche la raccomandazione della Commissione europea e l'opinione sul programma di stabilità 2023 sottolineano l'importanza di semplificare il sistema tributario, di aumentare gli incentivi al lavoro e di rafforzare la *compliance*, mantenendo la progressività del sistema. L'ultima vera riforma fiscale italiana risale agli anni Settanta: era calibrata sulle esigenze della società di allora,

Nel 1973 entrarono in vigore le disposizioni comuni in materia di accertamento, sulle agevolazioni tributarie e sulla riscossione delle imposte sul reddito, fino al complessivo riordino delle imposte sui redditi avvenuto con il testo unico del 1986. Da quel momento, si susseguirono diversi interventi di manutenzione: nel 1992 entrarono in vigore le disposizioni sul processo tributario e nel 1997 fu abrogata l'imposta locale Vennero poi introdotte alcune correzioni alla disciplina dell'IVA e venne anche riscritta quella relativa alle riorganizzazioni aziendali. Nel 2003-2004 ci furono interventi mirati

Complessivamente, parliamo di oltre 1.200 interventi in materia di imposte sui redditi e di oltre 500 in materia di IVA, che hanno fatto perdere coerenza e anche intellegibilità, prestando il fianco ad elusioni e facendo esplodere il numero dei contenziosi tributari, gestiti da una magistratura non dedicata, che ha visto approvata la necessaria riforma solo nel 2022.

Una svolta strutturale era quindi necessaria: durante la scorsa legislatura, il Governo Draghi e le Commissioni finanze di Camera e Senato hanno svolto un serio lavoro, che ha portato all'approvazione - in Consiglio dei ministri prima e alla Camera dei deputati poi - di un disegno di legge di delega fiscale. In questa riedizione del disegno di legge disegno di legge fiscale, molti dei princìpi di delega sono stati ripresi tali e quali: penso al principio di alleggerimento della pressione fiscale e di semplificazione della struttura dell'imposta, alla revisione e all'alleggerimento delle deduzioni e detrazioni d'imposta, alla revisione della tassazione dei redditi finanziari, con il conseguente superamento della suddivisione tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria. sulle attività produttive (IRAP) e al conseguente diverso finanziamento del sistema sanitario nazionale, con addizionali e sovraimposte, che dovrà essere attentamente studiato per non indebolire il già precario equilibrio della sanità italiana. Penso anche alla semplificazione della struttura dell'Ires, con il superamento delle variazioni fiscali e quindi l'avvicinamento del bilancio fiscale a quello civilistico. alla possibilità per gli autonomi di versare le imposte dirette mensilmente, abolendo così l'applicazione della ritenuta d'acconto, ed anche all'introduzione (IRI) per le società di persone, introducendo con questa nuova imposta proporzionale il superamento dell'attuale sistema di tassazione degli utili per trasparenza sui soci. È stata inoltre confermata la soppressione delle microtasse e confermata la priorità di un riordino di tutta la normativa tributaria dei testi unici. Quest'ultimo riordino è dettato dalla consapevolezza che l'Italia, secondo i dati della Banca mondiale, risulta essere 128° Paese al mondo quanto a semplicità fiscale. Anche in materia di riscossione, l'impostazione della delega fiscale del Governo Draghi viene mantenuta, ribadendo princìpi di delega quali l'orientamento al risultato nell'attività di riscossione, la simmetria degli interessi tra quelli che lo Stato applica e quelli dovuti ai contribuenti e il superamento della distinzione tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione. Resta prioritaria la più efficace gestione del magazzino fiscale, che oggi ha un controvalore di cartelle non riscosse pari a oltre 1.000 miliardi. Diverse dal Governo Draghi sono invece le modalità di prevenzione dell'elusione e

Per il sistema sanzionatorio è stato riproposto il criterio della proporzionalità, in linea con i meccanismi adottati, sia in sede Europea, sia in sede internazionale e come richiesto dalla Corte costituzionale. Quanto all'attuale sproporzione basti pensare, ad esempio, che in materia di IVA l'Italia applica sanzioni che oscillano dal 120 al 240 per cento, mentre in Europa ci si attesta sul 60 La proporzionalità e la certezza del diritto devono tornare a essere garantiti al contribuente, così come la piena applicazione dello statuto del contribuente, che nemmeno con questa occasione ha potuto assumere il rango costituzionale. Nella seconda parte della delega, dal punto di vista delle autonomie speciali è apprezzabile, ancorché riformulato, che il Governo in sede di conversione abbia recepito l'emendamento che prevede come, in sede di attuazione della delega fiscale, sia garantita l'invarianza del gettito spettante alle Regioni ad autonomia speciale e alle Province autonome, confermando lo strumento giuridico dell'intesa. Rispetto invece all'emendamento del Gruppo Per le Autonomie sulla clausola di salvaguardia, non è stato accolto in maniera integrale, ripiegando su una formulazione su una formulazione assai debole. Prendiamo comunque positivamente atto delle dichiarazioni e delle rassicurazioni del vice ministro Leo rispetto alle autonomie speciali e alle Province autonome di Trento e di Bolzano e agli aggiornamenti di cui da questo punto di vista si potrà tenere conto in sede di stesura del prossimo bilancio. In conclusione, da un lato vi è la necessità di avviare una transizione verso un sistema fiscale che favorisca la crescita economica, che rispetti il criterio dell'equità orizzontale, che riduca sensibilmente la pressione fiscale, nonché l'elusione e l'evasione fiscale e che sia più rispettoso dei rapporti tra fisco e contribuente; dall'altro, la realizzazione della riforma, con particolare riferimento alla razionalizzazione delle imposte, è subordinata alla disponibilità di risorse di cui, né nel DEF 2023, né nel rendiconto approvato la scorsa settimana, c'è conferma. Tale disponibilità va prioritariamente ricercata in una ricomposizione del prelievo, nel contrasto all'evasione fiscale e nella riduzione delle spese, perché la riforma dovrà realizzarsi nel rispetto della solidità dei conti pubblici e della sostenibilità del debito nel medio e lungo termine.

rappresentante del Governo, colleghi, il paradosso di questa discussione è che le forze politiche che hanno sostenuto il Governo Draghi, che è la matrice identificativa di questo disegno di legge lo rinnegano e si schierano addirittura con un atteggiamento contrario a tale disegno di legge. Le forze politiche che hanno assunto dal Governo Draghi le coordinate fondamentali di questo provvedimento

cui piace raccontare la verità ai cittadini e, se ci riusciamo, ci piace anche avere un minimo di coerenza rispetto all'impostazione dei governi che abbiamo sostenuto. Anzi, vorrei dire con precisione che noi abbiamo voluto noi abbiamo voluto quel Governo, mandando a casa il Governo Conte, e rivendichiamo la bontà di quella scelta. Ne rivendichiamo anche le battaglie più difficili, quelle che hanno aperto anche discussioni interne, per cercare di migliorare il fisco in questo Paese. È la ragione per la quale oggi noi ci schieriamo da una parte coerente: a favore di questo disegno di legge delega, consapevoli che nasce nell'impostazione dal Governo Draghi e lo dimostra - anche se magari non vorrà essere tirato in mezzo - la presenza del ministro Giorgetti. Non capiamo per quale motivo, da un lato, si voglia raccontare questo come un provvedimento che nasce solo dal Governo Meloni, ma non capiamo nemmeno per quale motivo chi stava dalla parte del Governo Draghi oggi rinneghi l'impostazione di questo disegno di legge

le forze dell'opposizione e gliene voglio dare atto, perché ha saputo ascoltare e lavorare con sapiente collaborazione. Per quanto riguarda la sottoscritta è la prima volta che collaboro con il vice ministro Leo. Siccome in questo Governo non è presente sempre una capacità una capacità di ascolto puntuale dell'opposizione, penso che oggi gliene dobbiamo dare atto *(Applausi)* e penso che anche il risultato del voto che portiamo sia, da questo punto di vista, giustamente il frutto di tale capacità di ascolto. Noi d'altronde, con grande serietà, abbiamo cercato di migliorare l'impostazione della legge delega. Abbiamo esteso le semplificazioni e il rafforzamento del sistema della riscossione nazionale anche ai sistemi di riscossione superando ripetizioni e offrendo ai Comuni una capacità operativa maggiore. Spesso sento parlare dei Comuni, ma il tema della riscossione nei Comuni piccoli è spesso un problema molto serio, perché si deve scegliere se internalizzare il servizio o esternalizzarlo, ma spesso non ci sono nemmeno le risorse umane sufficienti per fare un lavoro puntuale. Quindi, da questo punto di vista, siamo orgogliosi di aver avuto un occhio di riguardo in favore di quelle realtà, anche piccole, che faticano a recuperare risorse, a proposito di lotta all'evasione e a proposito di capacità di dare risposte a realtà territoriali piccole. Abbiamo precisato che nella proposta di concordato preventivo biennale, l'Agenzia delle entrate dovrà tenere conto del caso in cui il contribuente sia soggetto ISA, così così da definire i margini di discrezionalità che possono diventare vessatori per i contribuenti. Abbiamo chiesto una revisione e una razionalizzazione complessiva degli abbiamo chiesto l'introduzione del divieto per l'Agenzia dell'entrate di sanzionare il contribuente che aveva corretto una propria dichiarazione dei redditi sulla base di indicazioni elaborate dall'erario; abbiamo chiesto l'introduzione di un principio secondo cui, se c'è un processo penale che accerta determinati fatti di rilievo tributario, in caso di assoluzione del contribuente imputato,

chiesto un passo verso il federalismo fiscale, in un'ottica di modernizzazione del Paese, che rimane comunque un obiettivo centrale per noi. Ecco il modo e la postura con la quale ci siamo approcciati a un provvedimento il cui perimetro di fondo era stato costruito dal Governo Draghi, ma che necessitava di alcune correzioni. Tra queste correzioni il tema del prelievo forzoso, per evitare che questo Governo, dopo aver raccontato che non avrebbe mai messo le mani nelle tasche degli italiani, si approcciasse con una logica sbagliata anche a questo tema. Questo è il vero racconto di ciò che è avvenuto, il resto è propaganda e a noi non interessa. Rimane però un punto politico e lo dico al Governo in modo molto chiaro, ovviamente attraverso di lei, signora Presidente. Presidente. Si può anche riformare il fisco e fare in modo che sia più amico dei cittadini: lo si deve fare cercando di superare anche logiche politiche che sono figlie del passato. Mi diceva prima la collega Fregolent quanta difficoltà per liberi professionisti, avvocati e commercialisti dopo la fase del Covid, anche nella città dalla quale viene lei, a causa delle obiettive difficoltà economiche che il Paese ha vissuto, ma anche per l'appesantimento burocratico che queste categorie hanno subito.

non nel dire no alla legge delega sul fisco; occorre inchiodare il Governo attualmente in carica a ciò che è necessario fare in questo momento per aiutare il ceto medio. Abbiamo un'inflazione che cresce, abbiamo un aumento delle spese in tutte le direzioni. Questo Governo ha fatto i proclami sui tagli delle accise e poi le ha aumentate: questa è la verità dei fatti e non è possibile negarlo *(Applausi).* Allora dobbiamo chiedere di essere molto seri sulle questioni che interessano davvero la vita degli italiani. L'ho detto nei giorni scorsi e torno a ripeterlo anche oggi, non perché sia un mio assillo, ma perché lo ritengo il problema numero uno del Paese: occorrono interventi seri sul tema dei servizi e della sanità. Questo è il tema che abbiamo di fronte, quindi ben venga il fatto di intervenire con provvedimenti che ridisegnano il sistema, ma poi il cuore del problema lo avrete in autunno avrete in autunno ed è la legge di bilancio, la capacità di evitare che per i cittadini ci siano aumenti di tasse, il dare risposte serie sulle questioni delle accise, il fatto di continuare a sostenere l'economia e l'industria. Anche da questo punto di vista - perché poi si torna sempre lì - senza una crescita adeguata il Paese non potrà redistribuire nulla. In questo momento anche sul piano anche delle politiche industriali non vedo una capacità di visione lungimirante da parte del Governo. Noi, con grande serietà, oggi facciamo un atto di fiducia nei confronti di una revisione che ha obiettivamente dei pregi, anche delle ombre, ma tante luci

sostituire un'assenza di visione strategica sul Paese e una capacità di guardare agli italiani soprattutto con un occhio di riguardo e una capacità di recupero del potere d'acquisto da parte del ceto medio.

e senatrici, intervengo per fare una dichiarazione di voto sulla posizione di Forza Italia in merito alla delega fiscale di cui stiamo discutendo e che sarà un elemento innovativo per questo Paese, perché era era dagli anni Settanta che non si metteva a mano, se non attraverso una serie di interventi *spot* di superfetazione di norme, al sistema fiscale. Il disegno di legge al nostro esame è un tassello fondamentale del programma di Governo. Per Forza Italia si può certamente dire che la riforma fiscale è la stessa ragione sociale. Il presidente Berlusconi ha sempre avuto al centro della sua idea di Stato quella di un fisco amico del cittadino, a misura di impresa e a tutela del bene primario degli del bene primario degli italiani: la casa. Il suo *slogan* era - e continua ad essere, in quanto le sue idee continuano a vivere - meno tasse sulla casa, meno tasse su chi lavora e meno tasse sulle imprese. Questa riforma articola in modo molto netto un'idea di fisco a misura del cittadino e del contribuente. Meno tasse non significa, però, meno entrate fiscali, che sono necessarie e fondamentali per sostenere i servizi dello Stato a favore dei cittadini, vuol dire un carico fiscale più equo, che premia la crescita e la produttività, cioè un fisco che contribuisca alla prosperità delle famiglie, allo sviluppo delle imprese, alla creazione di posti di lavoro e all'espansione dell'economia e del benessere nazionali. Di conseguenza, insieme alla crescita del prodotto interno lordo, potrà realizzarsi anche una graduale riduzione della pressione fiscale, che rimane il nostro principale obiettivo. Nel merito del disegno legge, bisogna innanzitutto ricordare che questo è un collegato alla legge di bilancio 2023-2025. Questa circostanza comporta non solo che esso sia parte del programma di riforme del Governo, ma altresì che dai provvedimenti attutivi della delega, cioè gli appositi decreti delegati, siano attesi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica probabilmente già a partire dal 2024. Viene infatti rivisto il sistema tributario nel suo complesso, attraverso princìpi e criteri direttivi generali, stabilendo le modalità di coordinamento con la normativa vigente e individuando le norme da abrogare. Si tratta quindi di una delega che intende superare sia le riforme precedenti, sia la stratificazione normativa in materia fiscale che prosegue dagli anni Settanta. Il vero cambio di paradigma di questa riforma fiscale è nell'idea che lo Stato possa attuare accordi preventivi con i contribuenti sulla base dei quali programmare l'imposizione fiscale. Questo nuovo approccio, rivolto soprattutto alle categorie produttive, prevede un adempimento collaborativo che consente al contribuente di gestire, misurare e controllare il proprio rischio fiscale. Il rischio fiscale può essere certificato dai commercialisti e dai professionisti a questo abilitati e prevede sia una riduzione di due anni sui tempi di prescrizione degli accertamenti, sia l'esclusione delle sanzioni quindi è un grande vantaggio per la collettività. Per questa ragione vengono perfezionati e razionalizzati anche gli indici di affidabilità fiscale. Il risultato sarà attivato da intese tra i contribuenti e il fisco, finalizzate ad adottare delle proposte di tassazione possibile. Noi siamo felici che questi princìpi siano stati approvati dalla Commissione finanze del Senato, la quale mi onoro di rappresentare in qualità di Capogruppo del partito di Forza Italia

sullo stesso debito si duplicavano i pignoramenti. Questo ha segnato una nuova e concreta svolta rispetto alla tassazione del lavoro autonomo, ma bisogna rilevare che il Parlamento ha esaminato in modo ampio e completo tutti gli aspetti della riforma, avvalendosi dell'esperienza delle categorie professionali e imprenditoriali, che sono state ascoltate attentamente sia alla Camera che al Senato. La Camera in prima lettura ha modificato il testo del Governo, il Senato lo ha ulteriormente integrato e migliorato. Ora si prevede l'approvazione definitiva del disegno di legge prima della chiusura estiva, come ben sapete. I prossimi mesi serviranno quindi a scrivere i dettagli dei decreti previsti dalla delega. Certamente siamo convinti che si tratti di principi volti a introdurre un fisco più giusto, ma l'intenzione e gli effetti sono ovviamente anche quelli di limitare l'evasione e i contenziosi fiscali. Finora infatti l'accertamento e la repressione hanno dimostrato di non riuscire a generare nuove entrate consistenti, ma al contrario hanno creato presso l'Agenzia delle entrate un gigantesco magazzino di crediti non riscossi di circa 1.100 miliardi di euro. Siamo convinti che i princìpi generali cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega saranno largamente condivisi dai cittadini italiani, perché ormai è ineludibile mettere in campo un sistema fiscale capace di stimolare la crescita economica. È necessario, proprio attraverso il sistema fiscale, porre in atto tutti gli strumenti per agevolare la creazione di una famiglia, per favorire la natalità, per alleviare la disabilità. Pertanto era ed è fondamentale razionalizzare e semplificare l'intero sistema fiscale, facilitando un migliore rapporto tra cittadini e Stato. Cittadini e Stato devono stare sullo stesso piano e al cittadino devono essere dati gli strumenti e i tempi per difendere le proprie ragioni. È inoltre diventato irrimandabile il tema della riduzione della mole di adempimenti delle dichiarazioni e dei versamenti per i contribuenti.

Solo con un fisco più amico, prevedendo e limitando l'evasione, si può ridurre il carico fiscale medio sui cittadini. Rimane inalterato il criterio della progressività dell'imposizione fiscale: principio sancito dalla nostra Costituzione. In Senato è stata introdotta anche una nuova fiscalità degli enti territoriali, con un'attenzione particolare alle fonti di finanziamento dei Comuni e delle Regioni, in attuazione del cosiddetto federalismo fiscale. Gli enti del territorio devono poter programmare e gestire le proprie risorse con certezza, posto che sono i livelli di governo che devono dare le risposte più immediate ai cittadini attraverso i propri servizi. La delega prevede inoltre una graduale riduzione dell'Irap fino al suo completo superamento, mentre l'Ires, l'imposta sulle società, annuncia anche una riduzione di aliquota per le imprese che investono i propri utili o effettuano nuove assunzioni. Si tratta di un segnale, di un chiaro incentivo agli imprenditori ad investire i propri utili nella propria impresa attraverso dei premi evidenti alla crescita dimensionale aziendale e a chi crea posti di lavoro. Il fisco viene inoltre riformato anche rispetto agli aspetti internazionali e sovranazionali del sistema tributario, evitando forme di erosione e di elusione fiscale oggi consentite dall'applicazione di diverse discipline. Il fatto di avere collaborazione anche con il fisco di altre nazioni e creare un'omogeneità di trattamento è utile per evitare l'elusione fiscale. Al centro della riforma sta quindi il cittadino, che viene ad avere un ruolo paritario rispetto allo Stato, posto che è prevista anche la completa revisione dello statuto dei diritti del contribuente. Allo stesso tempo viene rinforzato l'obbligo di motivare e documentare gli atti impositivi e vengono valorizzati i princìpi di legittimo affidamento e di certezza del diritto. Proprio in questo senso è stato disciplinato anche l'istituto della consulenza giuridica, ben distinto dall'interpello, che avrà i propri presupposti, procedure ed effetti sugli atti fiscali. Viene inoltre istituita la nuova figura del garante nazionale del contribuente, operativa in ogni direzione delle entrate regionali e delle Province autonome. Proprio nel rispetto dei princìpi della progressività viene ridisegnata la revisione e la graduale riduzione dell'Irpef, l'imposta sui redditi delle persone a carico dei cittadini, verso una *no tax area* unica per le diverse categorie di contribuenti. La riforma mette inoltre mano al sistema delle agevolazioni, cosiddette spese fiscali, che prevede un articolato sistema di detrazioni e deduzioni. Questa verrà attuata con particolare attenzione alla composizione del nucleo familiare, alla tutela del bene casa, della salute, dell'istruzione e delle disabilità. Per quanto riguarda gli immobili, i redditi fabbricati vedono l'estensione della cedolare secca anche ai redditi da fabbricati adibiti ad uso diverso da quello abitativo, qualora il conduttore sia un esercente, un'attività di impresa o di arti o professioni. Sono previsti anche princìpi e criteri direttivi per i redditi di natura finanziaria, per i quali è prevista la creazione di un'unica categoria reddituale. Il valore di questi redditi viene determinato sulla base del principio di cassa, al fine di garantire la compensazione tra componenti positive e negative, limitando ovviamente gli spazi di elusione ed erosione dell'imposta. Sono previste forme di agevolazione e semplificazione sui rendimenti finanziari delle forme previdenziali complementari, che sono anche un importante forma di risparmio e per gli enti previdenziali privati. Viene inoltre prevista la possibilità di adottare una tassazione sostitutiva d'imposta sui redditi e l'addizionale applicabile ai redditi finanziari. È prevista infine la razionalizzazione delle aliquote IVA che grava sui consumi. L'obiettivo finale è arrivare a una codificazione, a una semplificazione a favore del contribuente di tutte le norme di carattere fiscale. Per concludere siamo in presenza di una riforma ben studiata e ben scritta che, oltre a segnare un nuovo rapporto tra cittadino e Stato, può segnare un punto di svolta per lo sviluppo economico del Paese. Una riforma che noi di Forza Italia voteremo convintamente e che dedichiamo al presidente Silvio Berlusconi, colui che per primo ha voluto fortemente un sistema fiscale basato sulla centralità e la premialità del contribuente.

quello della maggioranza non persegue la redistribuzione della ricchezza, non riduce di un euro le tasse sul lavoro e sulle imprese, non sostiene lo sviluppo economico e indebolisce lo stato sociale. Ringrazio comunque per l'impegno e la disponibilità profusa il vice ministro Leo. So che siamo lontani da quel tenore e da quello spirito dell'ultima vera riforma, la riforma Visentini del 1974. La vostra non è una riforma organica del fisco, ma un insieme caotico e confuso di misure *(Applausi)* che, nonostante le enunciazioni di principio, in realtà non farà non farà altro che rendere il nostro sistema tributario più complesso, frammentato, iniquo e non sostenibile. Diverse, pertanto, sono le contraddizioni e le ambiguità del disegno di legge in esame e proverò a sintetizzarne alcune. Viene enunciato il principio di equità orizzontale in base al quale, a parità di reddito, ognuno dovrebbe pagare le stesse imposte, ma introducete una serie di imposte sostitutive, andando a frammentare il sistema tributario con una serie di microimposte proporzionali, peraltro in presunta violazione del principio costituzionale della capacità contributiva. Il risultato sarà che forse ogni contribuente, in relazione alle diverse tipologie di reddito, pagherà un'imposta come capita. In questo modo accelerate la cosiddetta fuga dall'Irpef, con i conseguenti rischi inevitabili di sostenibilità del sistema fiscale. Viene poi enunciato il principio di progressività ed equità del sistema tributario, ma nei fatti la progressività diventa sempre più un miraggio e finisce per essere applicata solo ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, i soli che ormai sostengono il gettito Irpef. *(Applausi)*. La riforma fiscale quindi per tassare il lavoro e favorirà il ceto più ricco grazie alle molteplici *flat tax,* che risultano inique, irrealizzabili, insostenibili, tanto che da più parti ormai vengono definite *flop tax.*

lo stato sociale e anche gli investimenti, come peraltro avete già fatto nella legge di bilancio, escludendo i percettori del reddito di cittadinanza occupabili,

La stessa relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato ha già denunciato la mancata copertura finanziaria della sbandierata tassazione piatta sui premi di produttività e sulle altre indennità del lavoro. La riforma, inoltre, non sposta neanche di un euro la tassazione dai normali fattori della produzione, ovvero lavoro e imprese, alle nuove forme di ricchezza, quali quelle rinvenienti dall'economia digitale, dalle rendite finanziarie e dagli extraprofitti inaspettati legati ad eventi straordinari. Su questi tre temi abbiamo proposto una serie di emendamenti, come quello teso a realizzare una piattaforma unica del dato digitale, per arrivare ad una giusta tassazione dell'economia del *web,* nella consapevolezza che oggi lo sfruttamento dei dati digitali costituisce sempre più il nuovo petrolio da cui si generano ricchezze mai viste prima. Abbiamo anche proposto una tassazione progressiva sulle rendite finanziarie, inversamente proporzionale alla durata dell'investimento, in modo da contrastare la speculazione e favorire gli investimenti stabili. Abbiamo altresì proposto una tassazione strutturale degli extraprofitti imprevedibili ed emergenziali, in modo tale da destinare queste risorse ad affrontare le difficoltà e sostenere i cittadini in difficoltà. Nessuna di queste proposte è stata accolta dal Governo, che invece si è preoccupato bene di fare un altro regalo a quelle imprese energetiche che hanno fatto profitti, anzi extra-profitti, nel periodo dell'emergenza energetica. Oltre ad aver dimenticato il recupero del gettito fiscale di una norma scritta male durante il Governo Draghi, addirittura nel cosiddetto caldo avete fatto un altro regalo a queste imprese, perché avete rinviato la scadenza del pagamento del contributo di solidarietà sugli extra-profitti, che dovevano essere pagati entro il 30 giugno, spostandola entro il 30 novembre, senza interessi e sanzioni. Vi siete dimenticati degli alluvionati, visto che proprio oggi avete bocciato un emendamento, in cui avete negato la possibilità di rinviare le scadenze fiscali, così come non avete accettato la proposta dei dottori commercialisti, che sono in difficoltà, che vi hanno chiesto di spostare la scadenza dal 31 luglio al 30 agosto, come sempre è avvenuto, e non avete accettato questo emendamento Quindi, anche in questa occasione il Governo si conferma debole con i forti e forte con i deboli. In tema poi di equità, di redistribuzione e di riduzione della pressione fiscale, temi a voi sconosciuti, abbiamo proposto un innalzamento della *no tax area* per i redditi fino a 12.000 euro e una riduzione per sostenere gli aumenti salariali più bassi nelle grandi imprese, la cosiddetta norma Olivetti, volta a parametrare il salario più povero al salario del *manager* più alto in grado, ma anche questa, nel rapporto di uno a 50, ce l'avete bocciata. Considerate che oggi questo rapporto, in molte grandi aziende, anche italiane, arriva ad essere di uno a 600. Sul tema della semplificazione, abbiamo fatto una serie di proposte: anche qui fate una serie di reclami, ma senza concrete risposte in termini di scadenze fiscali e di recuperabilità delle detrazioni fiscali. Sul tema, abbiamo proposto per l'ennesima volta il *cashback* fiscale per favorire e semplificare la vita dei cittadini, ma anche questa proposta è stata bocciata. poi reso persino complessa l'unica tassa piatta esistente per le società di capitali, ovvero l'Ires, introducendo una sovraimposta in sostituzione dell'IRAP, che genererà ulteriori iniquità, perché verrà pagata solo dalle società di capitali, con conseguente aggravamento della pressione fiscale nei loro confronti. La complessità che persiste in questa proposta proposta di legge costringerà molti contribuenti a fare ricorso alle istanze di interpello: peccato che le avete rese a pagamento. Quindi, oltre ad un problema di iniquità, che poi produrrà tutta una serie di effetti sulla sostenibilità fiscale e sociale, vi è poi un altro tema che voglio evidenziare, quello della sostenibilità sociale minacciata dal decentramento della centralità fiscale alle Regioni, per effetto dell'autonomia differenziata. vorrei soffermarmi sul tema del contrasto all'evasione fiscale: onorevoli colleghi, parlate di pace fiscale, ma la vostra pace fiscale è solo per gli evasori. Non siete stati contenti degli oltre 11 condoni della legge di bilancio. In questa riforma, in questo disegno di legge delega, sono annoverati altri condoni. In particolare, viene introdotto lo scudo penale preventivo, legalizzando l'evasione per necessità e riconoscendo persino un abbuono economico per i salvati all'illegalità fiscale. Inoltre, ponete uno *stop* alle sanzioni penali tributarie connesse al reato di infedele dichiarazione per chi collabora e inventate l'evasione collaborativa. Infine, prevedete anche l'interruzione del procedimento tributario in caso di assoluzione in quello penale, cancellando quindi il principio del doppio binario e, a questo punto, riducendo il potere accertativo dell'Agenzia delle entrate, basato sulla presunzione semplice. Sono quindi ben 16 i condoni fiscali, perché oggi stesso la relatrice ha presentato l'ennesimo condono. Vado alle conclusioni, signor Presidente. L'unica vera riforma fiscale, tanto attesa dai cittadini, è quella che riduce le tasse. Voi questa promessa l'avete tradita per l'ennesima volta: avete avuto una grande occasione di ridurle con questa riforma, ma non le riducete. Per ridurre la pressione fiscale, occorre che tutti paghino le tasse, recuperandole da chi non le paga, scoraggiando l'evasione fiscale, colpendo i grandi capitali e tassando l'economia digitale e la speculazione economica e finanziaria.

di Rousseau: «La democrazia esiste laddove non c'è nessuno così ricco da comprare un altro e nessuno così povero da vendersi». Con questa riforma fiscale

Signor Presidente, colleghi senatrici, colleghi senatori, ovviamente la Lega voterà a favore di questa delega fiscale. Colgo innanzi tutto l'occasione per ringraziare il vice ministro Leo, il ministro Giorgetti, il sottosegretario Freni e tutti i membri della Commissione

Si è parlato molto della riforma fiscale, soprattutto in relazione alle aliquote Irpef e alle tasse alle imprese.

A cosa serve il fisco? Serve a incassare risorse dai cittadini per erogare servizi, e questa è la riscossione. Per farlo, però, serve anche calcolare quanto si deve pagare, e questo è l'accertamento. Ebbene, non funzionano né la riscossione né l'accertamento, ma questo non da adesso, bensì

oggi sono 1.153 miliardi. È aumentato enormemente, perché ogni anno aumentava con Governi di tutti i colori. Quindi, non vi è la volontà politica di non incassare le tasse *(Applausi).* Semplicemente, il sistema non funziona. Faccio un esempio per capirci, perché in questo magazzino c'è di tutto: ci sono le multe, come le famose buste verdi che abbiamo tutti; più

Peccato che, quando il contribuente fa ricorso, una volta su due vince, vale a dire che il 50 per cento delle volte ha ragione il cittadino e ha torto lo Stato.

lo Stato, non è stato in grado di incassare, quella cartella non esiste più. Qualcuno dirà che così non va bene, ma non funziona così: la cartella esattoriale è come il latte, dopo un po' semplicemente scade e la butti via

miliardi. L'operazione fa finalmente chiarezza, ma ciò vuol dire che tutti devono darsi da fare per essere più efficienti. Prendiamo il caso degli enti locali: se un ente locale non svaluta a bilancio le multe o la tassa sui rifiuti non incassabile, poi si trova con un buco di bilancio e questo alla fine non va bene, è polvere sotto il tappeto. Bisogna poi vedere che c'è una correlazione netta fra enti che vanno in predissesto e poi in dissesto: noi dobbiamo evitare questo. Non è un caso che, per esempio, abbiamo approvato due misure proprio su questi punti. Mi

Veniamo all'altro tema: l'accertamento. Abbiamo visto prima che l'attuale sistema non funziona. Per i lavoratori dipendenti - è chiaro l'abbiamo detto - è più semplice. Per i lavoratori dipendenti si va a dare una mano, per esempio detassando la tredicesima, poi abbassando le aliquote Irpef. Ma, sull'accertamento e su come si calcolano le imposte vi è un'enorme semplificazione: l'attuale sistema ha delle falle e allora noi cambiamo radicalmente. Facciamo una cosa semplice: ci fidiamo dei cittadini italiani. Dividiamo le aliquote in tre fasce. La prima fascia (*flat tax*) è fino a 85.000 euro: è facile, c'è la fattura elettronica, non scappa più niente, il fisco ha tutti i dati; fino a 85.000 euro il per cento: togli i costi, paghi quello e finisce lì, tutto semplice e veloce, tant'è che, da quando c'è, lo Stato incassa di più nell'ambito di questa fascia di cittadini.

Semplicemente noi vogliamo un sistema che, anziché pensare alle grida manzoniane che finora non hanno funzionato, e regole cervellotiche sempre più complicate che finora non hanno funzionato, pensiamo alla semplicità e alla fiducia. Questa è la riforma che vuole la Lega. Se ci sono semplicità e fiducia, lo Stato può e deve esigere rigore. Signor Presidente, noi pensiamo che il dibattito che è svolto nella giornata di oggi sia la sintesi più cruda e più vera di quanto siano lontane le posizioni sull'idea di fisco in Italia tra i principali Gruppi parlamentari e, quindi, tra i principali partiti. signor Presidente, che sia stata un'occasione persa. Pensiamo, ascoltando ora il presidente Garavaglia, che le parti siano molto lontane, e non tanto per la propaganda fisiologica che ogni Gruppo ha messo nel dibattito in Commissione e in Aula, ma proprio perché c'è una visione completamente diversa di qual è la funzione del fisco e di qual è la funzione dello Stato, quando deve tutelare quel recipiente di vimini. Signor ministro Giorgetti, *fiscus* era un recipiente di vimini dentro il quale c'erano monete dello Stato e, non monete dei singoli che pensano di tutelare se stessi indipendentemente dal ruolo che lo Stato riveste. *(Applausi)*. Quello che noi abbiamo sentito qui oggi dà il senso del fatto che questa delega fiscale racchiude tutti i motivi per cui destra e sinistra sono sedute dalla parte opposta di quest'Aula. Abbiamo due visioni diverse dopo questo dibattito inconciliabile. Voglio ricordare sommessamente alla senatrice Paita, che addirittura ha scomodato Draghi.

il sacrificio che il fisco deve cagionare deve essere uguale per ogni contribuente, perché questo è scolpito nella nostra Costituzione. Il fisco deve cagionare il medesimo sacrificio ad ogni contribuente, che non è la *flat tax*. Io non penso che al presidente Draghi potesse mai venire in mente una frase infelice come «pizzo di Stato», senatrice Paita. *(Applausi)*. Noi non c'eravamo non c'eravamo con questo concetto di fisco. E voglio dirlo al presidente Garavaglia, che è firmatario dei principali emendamenti che hanno portato questa delega ad essere, più che una delega fiscale - e mi dispiace perché riconosco

che l'Agenzia delle entrate sia non un pezzo dello Stato, ma un nemico dello Stato e dei cittadini italiani. *(Applausi)*. È andata in onda questa roba in Commissione finanze.

al tempo della società digitale, al tempo dell'intelligenza artificiale, al tempo del mondo aperto e senza confini, al tempo in cui l'Europa fa fatica a far le battaglie contro alcuni paradisi fiscali (cosa che noi dovremmo fare e pretendere). dovremmo fare e pretendere). Anziché questo, che cosa abbiamo fatto? In pochi giorni - e sottolineo pochi giorni - si è rotto, signor Ministro dell'economia, il rapporto di fiducia tra maggioranza e opposizione. Quando si fa un patto politico e si dice che la delega fiscale si tratta nei due rami del Parlamento nello stesso modo, con gli stessi tempi e si dividono le parti della delega fiscale in maniera uguale, se poi però viene tradito perché la delega resta tre mesi a Montecitorio e due settimane - solo grazie alla mediazione della Presidenza altrimenti sarebbe rimasta qui quattro giorni è evidente che vengono meno le ragioni che portano i Gruppi parlamentari di opposizione a fidarsi non del merito, ma del metodo. E quando viene meno questo, diventa difficile confrontarsi poi nel merito. andare su aspetti che sono fondamentali per noi. Penso che mai come in questa vicenda - ed è del motivo per il quale voteremo contro questa delega al Governo al Governo - il Governo ha strizzato l'occhio a quelli che vengono chiamati con benevolenza "tartassati", che ma in realtà sono furbetti.

le cose che ha anticipato il vice *premier* Salvini - lo dico soprattutto ai colleghi della prima forza politica di maggioranza, Fratelli d'Italia - sono tutte state trasformate in emendamenti che sono passati. Lo aveva anticipato con due o tre settimane di anticipo. Addirittura la delega era a Montecitorio quando il Vice Presidente del Consiglio aveva anticipato alcune misure. Vogliamo ricordarvi che, se alla fine di questo percorso ad un certo punto le risorse inevitabilmente verranno meno, a pagare non saranno i ricchi. E lo dico al senatore Orsomarso con il quale abbiamo condiviso una parte consistente del confronto. I ricchi possono pagarsi i servizi quando e come vogliono. Noi abbiamo detto più volte che avremmo dato la nostra disponibilità a entrare nel merito di una mediazione che doveva costruire un ponte - quello vero, non il ponte sullo Stretto - tra la delega fiscale e e l'autonomia differenziata. Ci avete detto di no. Ci avete detto che non era possibile. Ci avete detto addirittura - è l'ultimo passaggio andato in scena in Aula durante le dichiarazioni a margine degli emendamenti - che questo passaggio non era possibile perché, in realtà, non ci sono le condizioni per garantire sul disegno di legge delega e sull'autonomia

di *back office* nel nostro Parlamento e ci riesce anche bene, ma questo è il Parlamento e lei in questo momento è componente autorevole del Governo. Io le voglio sconsigliare, a nome del Gruppo Partito Democratico, di continuare a fare *mobbing* nei confronti dei Presidenti di Commissione, perché a un certo punto finisce anche la pazienza dei senatori. Le consigliamo di fare con correttezza il suo lavoro e poi di confrontarsi in ogni Commissione - come è giusto che sia - sul merito. Abbiamo tentato di costruirlo, questo ponte, signor Presidente, ma non ci siamo riusciti

signor Ministro dell'economia, che non aumentasse la pressione fiscale attraverso i tributi regionali per coprire trasporto pubblico locale, scuola, sanità e assistenza. E, se questo dovesse accadere, sarà un tradimento all'unità nazionale. *(Applausi)*. avete respinto l'emendamento che chiedeva semplicemente il rispetto di un principio, e cioè che nella delega fiscale ci fosse la certezza dell'impegno del Governo a istituire un fondo di perequazione che finanziasse dal centro i livelli essenziali delle prestazioni. È arrivato un no secco, immotivato e incomprensibile che aumenterà la divisione nel Paese non solo tra Nord e Sud, ma anche tra le aree più ricche e le aree interne, tra le aree più sviluppate che hanno più servizi e le aree di montagna. E il costo lo pagheremo tutti, perché in quelle aree vivono 12 milioni di italiani che non hanno meno diritti di chi vive nelle aree più sviluppate e più ricche del Paese. *(Applausi)*. in conclusione, sulla pace fiscale presunta abbiamo espresso il nostro giudizio di netta contrarietà e lo abbiamo fatto sapendo che sullo sfondo

oltre alle italiane e agli italiani di cui vi siete occupati, per la verità una minoranza, ci sono 16 milioni di pensionati che non avranno alcun beneficio da questa riforma fiscale. Ci sono 18 milioni di lavoratori dipendenti che ogni giorno contribuiscono ai servizi sociali di questo Paese. Ci sono gli autonomi, tra quei sette milioni, presidente Garavaglia, che, quando arriva quella busta verde, pagano puntualmente e non chiedono né di rottamarla, né di prendere tempo. *(Applausi)*. Ci sono tanti imprenditori che non hanno paradisi fiscali, che investono, pagano le imposte puntualmente e chiedono al Governo solo servizi pubblici migliori.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge delega per la riforma fiscale è uno dei provvedimenti senza dubbio più importanti del Governo Meloni, probabilmente dell'intera legislatura. Il testo che ci accingiamo a votare rappresenta, infatti, un caposaldo imprescindibile dell'azione del Governo, finalizzato a sostenere il sistema Paese, le famiglie e le imprese attraverso una riduzione degli adempimenti fiscali e delle aliquote dell'Irpef e dell'Ires, il superamento dell'IRAP e la revisione degli attuali 226 crediti d'imposta. Il lavoro svolto in prima lettura dai colleghi della Camera dei deputati e successivamente, in queste settimane, al Senato, rappresenta un risultato ambizioso che ha contribuito a migliorare ulteriormente il testo approvato lo scorso marzo dal Consiglio dei ministri.

Sono passati cinquanta anni. L'ultima legge risale al 1971, periodo in cui - come ha spesso ricordato il vice ministro professor Leo l'impostazione normativa adottata dal legislatore fiscale era contemplata sulla base di un codice civile che dettava poche regole, privo di un organismo italiano di contabilità. anni - grazie a questo Governo e a questa maggioranza, finalmente si mette mano ad un impianto normativo ormai vecchio, che ad oggi - senatore Menia - non può più evidentemente soddisfare le esigenze dei cittadini e dello Stato che col tempo sono palesemente cambiate. Ci troviamo di fronte a una svolta necessaria per il Paese, promessa fatta agli elettori che realizziamo solo dopo pochi mesi dall'insediamento del Governo Meloni *(Applausi)*, con il lavoro fattivo del Parlamento. sulla questione fisco abbiamo assistito a molti, moltissimi proclami, ma a pochi fatti; ogni Governo che ha preceduto questo Esecutivo ha proclamato grandi iniziative e un'infinità di dati, numeri e parole, alle quali quasi mai sono seguiti fatti. oggi abbiamo dei fatti di cui parlare. Oggi possiamo affermare che si è fatto un ottimo lavoro, una riforma fiscale e nuove regole per un fisco più semplice, sensato e in grado di garantire il funzionamento della macchina statale, senza indebolire le imprese e il sistema produttivo, e soprattutto che vede il contribuente come soggetto attivo e non vessato. Questo è il fisco che delinea la legge delega Vediamo però analiticamente quali saranno in maniera concreta, tangibile e reale le misure che da decenni le famiglie e le imprese italiane attendono innanzitutto attraverso la riduzione in maniera generalizzata del prelievo che grava su di loro, in un'ottica di semplificazione e di razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Le nuove regole vanno nella direzione di semplificare e ridurre la pressione fiscale, favorire investimenti e assunzioni, instaurare un rapporto tra contribuenti e amministrazione finanziaria nella logica di un dialogo mirato tra le parti, secondo le esigenze dei cittadini e delle imprese. L'attuale ordinamento fiscale non è certo una novità: è tra più complicati del mondo e non lo dice solo la Banca mondiale, ma lo dicono i cittadini e le imprese che dovrebbero occuparsi dei loro *core business* e non invece dei continui, ripetuti e infiniti adempimenti burocratici e fiscali. Era pertanto assolutamente necessario dopo decenni fare un po' di ordine, razionalizzare, accorpare e rendere più leggibile e comprensibile l'intricato sistema tributario italiano. Questo è il punto di partenza che ha voluto il Governo Meloni e in particolare il vice ministro Leo, che ringrazio così come hanno fatto tutti quanti i colleghi che mi hanno preceduto riorganizzare l'intero impianto delle norme tributarie del Paese, per arrivare finalmente anche a una diversa visione del rapporto tra fisco e contribuente. È stato rivisto anche l'intero sistema sanzionatorio con la riduzione delle pene pecuniarie e tributarie per allinearle agli *standard* di altri Paesi europei, con interventi mirati anche sul fronte del contrasto all'evasione i cui numeri sono allarmanti. Abbiamo ancora una *tax gap* che va dai 75 ai 100 miliardi di euro, che impongono di non abbassare la guardia. Come richiesto anche dall'OCSE, il disegno di legge delega interviene attraverso il concordato preventivo biennale con una sorta di patto

ma accordi preventivi per migliorare il rapporto tra il cittadino e il fisco. Il principio da cui siamo partiti per impostare la delega è che non esiste un occhio di riguardo per un comparto piuttosto che per un altro, che si tratti lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di lavoro d'impresa. L'obiettivo della diminuzione complessiva del carico fiscale che questo Governo di centrodestra finalmente realizzerà è sempre perseguito tenendo a mente gli equilibri di finanza pubblica da preservare. Con questa riforma fiscale il sistema diventerà più europeo, a differenza della cosiddetta controriforma presentata dai colleghi della sinistra, che prevede più tasse per tutti, per i redditi impresa e del lavoro.

un fisco più equo, meno ostile verso i cittadini e meno opprimente per le imprese e così è fatto. *(Applausi)*. La riforma fiscale è la fotografia di questo Esecutivo, il risultato di una visione economica e sociale che ha cominciato a dare i suoi frutti già con l'approvazione della legge di bilancio,

Nonostante il periodo particolarmente difficile per l'Europa, con l'inflazione che avanza e l'economia globale che frena, l'Italia cresce più di Francia e Germania e un dato del genere non si vedeva da decenni. Lo *spread,* cavallo di battaglia della sinistra, dell'opposizione - ovviamente solo quando è all'opposizione - oggi oggettivamente non desta preoccupazione: non a caso, la fiducia di famiglie e imprese verso questo Esecutivo è fortemente in aumento; i titoli di Stato sono una fonte di risparmio e di investimento; le famiglie hanno ripreso a credere nel futuro della nostra Nazione, investendo i loro risparmi. *(Applausi).* Questo, colleghi, avviene solo grazie al Governo Meloni. Le opposizioni puntavano ad un altro caso *spread,* al giudizio negativo delle agenzie di *rating,* al fallimento delle nostre iniziative, al blocco delle rate del PNRR. chi non ha idee cerca di farsi spazio screditando il lavoro degli altri, ma gli italiani sanno bene a chi hanno affidato il loro futuro. Questa è la differenza: c'è chi tifa per il Paese e chi non lo fa. Noi tifiamo per l'Italia. In questi mesi tutti gli sforzi sono stati concentrati nel restituire credibilità e solidità ad una Nazione che per anni è stata bistrattata; con i Governi precedenti per molto tempo si è navigato a vista, ma finalmente ora esiste una rotta che non si lascia ingannare dalle luci incerte di navi lontane che passano, ma che, attraverso la forza delle nostre idee, ci porterà verso mari sicuri. Questa è la dimostrazione che, se l'Italia è governata con consapevolezza, può ritornare ad essere la grande Nazione che è sempre stata. Per questi motivi sono onorato di poter annunciare convintamente il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. Avanti tutta!

La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che la discussione generale del decreto-legge concernente organizzazione della pubblica amministrazione,

Come già preannunciato, seguirà la già annunciata posizione della questione di fiducia da parte del Governo sul testo approvato dalla Camera dei deputati, con dibattito limitato alle sole dichiarazioni di voto. Seguirà la chiama, presumibilmente intorno alle ore 12. Restano confermati gli altri argomenti già previsti dal calendario, vale a dire l'esame del decreto-legge concernente la tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica

anche in precedenza, in relazione a situazioni di urgenza connesse con le materie di propria competenza. L'Assemblea tornerà a riunirsi martedì 5 settembre, alle ore 16,30, per la discussione generale di ratifiche di accordi internazionali ed eventuale seguito di argomenti non conclusi, con votazioni a partire dalla seduta di mercoledì 6 settembre.

un'esperienza che mi ha toccato profondamente, portandomi a riflettere sulla complessità del sistema carcerario e sulla sua effettiva funzione di preparazione al reinserimento sociale. Durante gli incontri con i detenuti ho avuto modo di ascoltare le loro storie, i loro rimpianti, le loro speranze. Mi hanno aperto il loro cuore con una sincerità disarmante, mettendo in luce la complessità delle loro vicende personali, fatte spesso di un passato difficile e di scelte sbagliate, a causa di circostanze avverse o di mancanza di opportunità. Sono soprattutto uomini giovani e meno giovani animati da un profondo desiderio di redenzione e di una seconda possibilità, intenti a fare progressi significativi nel percorso di recupero. Le visite nelle carceri mi hanno spinto a riflettere sul ruolo del sistema giudiziario e sulla necessità di promuovere una giustizia equa e proporzionata, che sappia anche tutelare i diritti dei detenuti. Il carcere racchiude in sé un duplice mandato: quello della custodia certo, ma soprattutto quello della rieducazione come opportunità sia per la riabilitazione e il reinserimento, sia per la stessa messa in sicurezza della nostra società. Mi chiedo: stiamo facendo abbastanza per offrire effettivamente una seconda possibilità ai detenuti italiani? La risposta è no. Non nascondo l'emozione che ho provato ascoltando la storia di un uomo condannato per reati secondari, che desiderava assistere alla comunione del proprio figlio ed era in attesa di un permesso che stentava ad arrivare, perché mancava il magistrato di sorveglianza. Onorevoli colleghi e colleghe, vi è una carenza di magistrati che pregiudica qualsiasi risposta alle esigenze e alle domande dei soggetti sottoposti a misure detentive e ne rallenta il percorso riabilitativo, lasciandoli spesso intrappolati nel circuito della devianza. Inoltre, viene disattesa l'applicazione delle misure alternative di detenzione, differenziate in base alla tipologia di reato commesso, fondamentale per l'attivazione di percorsi concreti di risocializzazione. Gli stessi permessi sono parte integrante del programma di trattamento dei detenuti, perché consentono di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro, come espressamente rimarcato dalla Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati. Per questo motivo ritengo che il Ministro della giustizia abbia il dovere politico e morale di stanziare fondi aggiuntivi già dalla prossima legge di bilancio per incrementare gli organici dei magistrati di sorveglianza, così da tutelare i diritti dei detenuti e garantire un clima più sereno negli istituti di detenzione. Sia chiaro: non è una questione di bandiera politica, ma di salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo, una sfida a cui questo Governo di centrodestra deve dare risposte concrete in tempi rapidi.

per ricordare una delle più orrende stragi che hanno insanguinato l'Italia e che provocò 85 morti e 200 feriti, persone normali di un'Italia quotidiana che ricordiamo tutti con dolore e affetto. Un ricordo personale. Tra i morti c'era anche un ragazzo di Terni, aveva ventiquattro anni, era laureato al DAMS e aspettava un treno: Sergio Secci, un carissimo amico, viaggi e vacanze insieme, sogni condivisi di ragazzi, sogni che Sergio lasciò lì, insieme alla sua vita. Tanti, troppi sono stati in questi anni depistaggi e complicità, però molte verità giudiziarie sono state raggiunte. Ad oggi sono stati condannati in via definitiva come esecutori materiali i terroristi neofascisti del NAR Fioravanti, Mambro, Luigi Ciavardini e, con altra sentenza precedente, un altro esponente nero come Gilberto Cavallini. Condannati definitivamente per attività di depistaggio sono stati il capo della P2 Gelli, il faccendiere Pazienza e ufficiali dei servizi segreti. Recentemente la corte d'assise di Bologna ha condannato all'ergastolo un altro neofascista, Paolo Bellini, considerato tra i mandanti. La strage di Bologna fu compiuta dentro una strategia di destabilizzazione della democrazia, con reti di complicità interne e internazionali, con massonerie e perfino pezzi dello Stato. Era la strategia della tensione, inaugurata il 12 dicembre 1969 con piazza Fontana, poi con piazza della Loggia e l'Italicus. I Gelli e gli Ortolani furono attori fondamentali di questa strategia nera ed eversiva. Questa mattina a Bologna, insieme al senatore Bazoli, eravamo alla manifestazione e lì i familiari e il loro presidente Bolognesi hanno chiesto di nuovo piena affermazione di giustizia e verità, senza vecchi e nuovi depistaggi. Su tutte è risuonata la voce del presidente Mattarella, che ha parlato di matrice neofascista e di ignobili depistaggi. Lo stesso ha detto il presidente della Camera Fontana e anche al presidente del Senato La Russa

proprio perché i Presidenti delle due Camere hanno pronunciato parole appropriate, esprimiamo sconcerto per il silenzio della Presidente del Consiglio, che non ha voluto, saputo, potuto pronunciarle, quelle parole: la strage di Bologna fu una strage neofascista. Sarà per questo che anche altri Ministri che, come Piantedosi, pure stavano a Bologna, sono stati silenti e reticenti. È molto grave per noi che la maggioranza alla Camera abbia votato una mozione anch'essa omissiva e reticente e di fatto depistante, respingendo quella del PD e di altre forze che chiedevano una cosa: si lascino lavorare uffici giudiziari nelle condizioni di autonomia totale, in modo da pronunciare sentenze definitive senza ingerenze, come per esempio le immancabili, inconsistenti piste palestinesi o con improbabili Commissioni di inchiesta parlamentari che sembrano fatte apposta per depistare. Aggiungo un'ultima cosa. Per noi non può e non deve essere permesso a nessuno di occultare responsabilità, riscrivendo persino la storia, sia quella sulla strage di Bologna che quella sulla strage di Ustica. Questo Paese ha già ha già pagato troppo con le stragi e nessuno può pensare di colpirlo ancora al cuore: sarebbe come spargere sale su ferite aperte che possono essere rimarginate solo con quelle due parole risuonate questa mattina alle 10,25 davanti alla stazione di Bologna: verità e giustizia.